391-*ter *e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del* web *e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale***

Tale questione darà origine, a nostro avviso e come abbiamo potuto constatare nel corso dell'esame in Commissione, a non pochi problemi dal punto di vista della successione delle norme nel tempo, essendo essa questione amministrativa o questione penale. Al di là di tutto, il decreto-legge tratta il tema dell'immigrazione in connessione con una pluralità di altri temi che assumono particolare rilevanza: il diritto costituzionale, il diritto internazionale e il diritto comunitario. Nella relazione illustrativa si specifica che l'intervento si rende necessario per rimodulare alcuni profili che tengono aperti taluni aspetti e principi costituzionali. Alla Camera sono state approvate ulteriori modifiche rispetto al testo originario del decreto con la novella dell'articolo 5 - testo unico sull'immigrazione - che ha ulteriormente allargato gli ambiti di applicazione di alcune norme, sia dal punto temporale che territoriale.

In altri termini, nel decreto-legge vi è un'affermazione apodittica sulla necessità di urgenza dell'intervento normativo,

lo strumento della decretazione d'urgenza è per sua natura strumento eccezionale e temporaneo e soprattutto non ripetibile. È evidente che interventi così immediati a breve distanza di tempo incidono non solo sull'articolo 77 della Costituzione, sotto il profilo della tenuta della necessità e dell'urgenza, ma anche sotto il profilo dell'articolo 70 della Costituzione, ovvero di un possibile sbilanciamento degli interventi normativi, dal momento che in questo caso il Governo prevale sulla funzione paritaria e bicamerale dell'iniziativa legislativa, che appartiene ai due rami del Parlamento.

il riferimento alla disciplina in materia di immigrazione, derivante dalla necessità di modificare i precedenti decreti Salvini, e ci troviamo davanti ad un provvedimento che abbraccia norme penali, introduce nuove sanzioni

Vi è sul punto la sentenza n. 22 del 2012, con cui la Corte ha ritenuto illegittimo il decreto-legge, se il suo contenuto non rispetta il vincolo dell'omogeneità. Si richiama una fonte di rango non costituzionale, ma pur sempre un atto avente forza di legge, ovvero l'articolo 15

l'intervento recente della Corte costituzionale, con la sentenza n. 247 del 4 dicembre 2019, in cui si è affermato che l'inserimento di norme eterogenee,

Grazie,

e non coerente e conforme ai principi e ai pronunciamenti più recenti della Corte, e per tale ragione insistiamo perché siano considerato i profili di dubbia legittimità dal punto di vista della tenuta costituzionale, sia in violazione dell'articolo 77, secondo comma della Costituzione, sia per quello sbilanciamento della funzione legislativa, indicata nell'articolo 70, che assegna condizioni paritarie, nell'esercizio della funzione legislativa, alle Camere.

Vorrei richiamare alcuni punti del testo uscito dalla Camera, che ha modificato il decreto-legge originario, in particolare con riferimento all'articolo 1, comma 1, recante disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera. Si è intervenuti sulla disposizione relativa al DPCM che stabilisce annualmente i flussi di ingresso stranieri. A seguito delle modifiche apportate si prevede che, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri possa provvedere in via transitoria Grazie, disciplina sostituisce quella introdotta dal Decreto "sicurezza bis" disponendo che il provvedimento di limitazione o divieto possa riguardare il transito e la sosta delle navi, senza più fare riferimento all'ingresso; È disposta l'esclusione per le operazioni di soccorso immediatamente comunicata al centro di coordinamento competente allo Stato di bandiera. Inoltre, si prevede, come ho detto prima - insisto su questo punto - l'abrogazione della sanzione amministrativa del divieto di ingresso nelle acque territoriali. Abbiamo cercato di dare una panoramica il più possibile esaustiva ed esauriente dei provvedimenti affetti da illegittimità costituzionale o quantomeno richiedono una valutazione, un esame pregiudiziale e impediscono l'esame nel merito del provvedimento. Vorrei ricordarvi anche l'uso strumentale che la maggioranza ha fatto di questi decreti-legge, dato il arrivando all'ultimo momento alla questione di fiducia, che viene di fatto posta a scatola chiusa, dopo pochi giorni di esame da parte del Senato, precludendo ulteriormente l'esercizio dell'attività legislativa e il controllo - da parte del Parlamento - sull'attività svolta svolta dal Governo. A nostro avviso, quindi, non ci sono requisiti di necessità e urgenza; a nostro avviso viene violato indirettamente l'articolo 70. Richiamo la Presidenza del Senato, come ha fatto l'altro giorno in modo molto chiaro il presidente Casellati, Signor Presidente, cari colleghi, condivido le osservazioni svolte poco fa dal collega Dal Mas e vorrei ricordare a quest'Assemblea così distratta che la nostra Costituzione, all'articolo 77, assegna al Governo il potere di intervenire, certo, con decreti-legge, ma soltanto in casi straordinari - e sottolineo la parola «straordinari» di necessità e urgenza. Un caso straordinario è un fatto eccezionale, che impone in modo inevitabile e

Già il fatto che per un anno e oltre si annunci un decreto-legge significa che non è più eccezionale né urgente. in materia di immigrazione, come se l'immigrazione fosse un fatto nuovo, sconosciuto, sul quale non sia intervenuta a tamburo battente una legislazione per molti anni, in ultimo quella del 2018 che voi, maggioranza e Governo, con il provvedimento in discussione volete stravolgere. In realtà, signor Presidente, non c'è nessun fatto eccezionale purtroppo, non c'è nessuna necessità e non c'è nessuna urgenza. L'unica urgenza che avete voi del Governo e della maggioranza è portare a termine ancora una volta il vostro disegno ideologico immigrazionista:

i disperati di tutto il mondo ricevano un messaggio chiaro e preciso dall'Italia: venite quanti più potete qua, siete accolti all'infinito. Questo è il messaggio che voi mandate con questo decreto-legge che, cari colleghi, palesemente incostituzionale perché, come sottolineava prima anche il collega Dal Mas, manca nel modo più assoluto

secondo la quale le norme contenute nel decreto-legge devono possedere un'intrinseca coerenza dal punto di vista oggettivo e materiale, ovvero funzionale e finalistico. L'urgente necessità di provvedere può così riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate o dall'intento di fronteggiare situazioni complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti a materie diverse, ma attenzione - indirizzate all'unico scopo di approvare rimedi urgenti. Nella comunanza di oggetto o finalità delle norme si caratterizza l'omogeneità del contenuto del decreto imposta dall'articolo 77 della Costituzione, che riferisce i presupposti della decretazione d'urgenza all'atto nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo. Conclude la Corte: in mancanza di omogeneità, il decreto-legge decadrebbe in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale. Ed è esattamente quanto succede con questo decreto-legge, perché, come ricordava anche il collega Dal Mas, è vero che dall'articolo 1 all'articolo 6 parliamo di immigrazione, ma l'articolo 7 modifica l'articolo 131-*bis* del codice penale; l'articolo 8 modifica l'articolo 391-*bis* del codice penale; l'articolo 9 introduce un nuovo articolo nel codice penale; l'articolo 10 modifica addirittura l'articolo 588 del codice penale in materia di rissa. L'articolo 11, in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici di chi abbia denunce... mi pare che fortunatamente non sia successo niente.

senatore Questore De Poli mi fa presente di avvisare i colleghi che siedono sulle tribune di non appoggiarsi alle cosiddette balconate

che l'articolo 11 del decreto-legge in discussione interviene in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici di chi abbia denunce o condanne per spaccio di droga o per reati commessi in occasione di gravi disordini. L'articolo 12 interviene in materia di contrasto al traffico di stupefacenti via Internet. L'articolo 13 addirittura interviene in materia di Garante nazionale dei detenuti. Si tratta di norme tra loro assolutamente Allora ci si chiede: quale può essere la finalità che accomuna tutte queste norme? Verrebbe da pensare che davvero, secondo voi, l'immigrazione crea gravi problemi in materia di spaccio di droga e in materia di sicurezza; questo potrebbe essere l'unico filo conduttore che accomuna tutte queste norme. Ma poiché la maggioranza e il Governo hanno sempre negato questa evidenza, allora bisogna concludere che non c'è alcun filo che accomuna tutte queste norme. Per rendermene conto sono andato a leggere il preambolo del decreto-legge. Come voi tutti sapete, colleghi, l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 al comma 1 impone

verificato se nel preambolo sono indicate le circostanze straordinarie di necessità e urgenza che ne giustificano l'adozione? Qualcuno di voi ha letto il preambolo? Cari colleghi che mi date le spalle mentre intervengo, cari Capigruppo della maggioranza che continuate a parlare dandomi le spalle mentre intervengo, avete letto il preambolo del decreto-legge? Avete verificato se nel preambolo sono indicate le circostanze straordinarie di necessità e urgenza che ne giustificano l'adozione? Lo avete letto? Io l'ho fatto e non c'è nulla. Vi faccio solo un esempio: modificate cinque articoli del codice penale. Come lo giustificate nel preambolo? Ve lo posso leggere? Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale. Questa è la giustificazione che, secondo voi, dovrebbe soddisfare il requisito indicato nell'articolo 15 della legge n.

incostituzionale e che, quindi, oggi si accolga la nostra pregiudiziale per chiudere qui l'esame di materie che richiederebbero ben altro approfondimento, ben altro dibattito e ben altra discussione rispetto ai pochi minuti che ci vengono concessi per esaminare questioni così importanti. *(Applausi)*.

in Aula con il casco e ovviamente con la necessaria mascherina. con un telefono in mano che sporge oltre la balaustra e l'altro ce l'ha in mano. Io credo che sia una recidiva quella che sta accadendo e richiedo un richiamo formale.

possibilmente anche capirla. Se, infatti, uno lo avesse fatto, apparirebbe immediatamente non necessario, urgente e straordinario il provvedimento al nostro esame. Partiamo dal primo requisito che dovrebbe avere un decreto-legge, ovvero - è la giurisprudenza della Corte che lo dice - il criterio della omogeneità. Non sto a ripetere quanto hanno detto i nostri colleghi prima. Se uno legge il titolo, vede che l'omogeneità c'entra come i cavoli a merenda rispetto ai contenuti di questo provvedimento e giustamente il Presidente del Senato l'ha assegnato alla 1a e alla 2a Commissione. Altrettanto giustamente il Presidente della 2a commissione ha chiesto che venisse assegnato anche alla propria Commissione per l'esame C'è stata una grossa polemica da parte della maggioranza rispetto a queste decisioni. La polemica è proseguita anche in Commissione, dove si è arrivati ad accusare il presidente Ostellari di aver mentito rispetto alle decisioni assunte. Qualcuno ha parlato di un falso in atto pubblico nel verbale della 2a Commissione. Ringrazio la senatrice Evangelista, che è intervenuta dicendo che il verbale era corretto e che il comportamento tenuto dal presidente Ostellari era assolutamente rispettoso di quello che era accaduto in Commissione.

Oltre a questo, vorrei ricordare a chi se lo è dimenticato che questo decreto modifica, nella parte prevalente, il decreto-legge Salvini 2. Nell'esame alla Camera dei deputati il presidente Fico ha assegnato il provvedimento alla I e alla II Commissione e nessuno ha detto niente. *(Applausi)*. fatta alla Camera dei deputati, è l'operazione di Fico e, quando viene fatta al Senato invece - non dico una parolaccia - è un'altra cosa, che ricorda il nome del Presidente della Camera. È la cosa più giusta, punto

I tre rilievi che fa riguardano gli aspetti sanzionatori e quindi il capitolo della giustizia. È il caso di citarli: parla delle sanzioni amministrative per il divieto di ingresso delle navi, navi, del rispetto dei vincoli internazionali e della norma relativa all'oltraggio a pubblico ufficiale. Tutto il resto che ci avete messo dentro non c'entra assolutamente niente.

Dov'era finito quel decreto-legge? Lo hanno tenuto nel cassetto per il salvo intese, per cui litigano su tutto, oppure addirittura qualcuno ci ha pensato sedici giorni prima di firmarlo e mandarlo alle Camere?

dichiarazioni degli esponenti della sinistra, dal primo giorno e tutti i giorni, la prima cosa necessaria e urgente da fare per il Paese era abolire i decreti-legge Salvini. Qualcuno può pensarla in quella maniera, peccato che fossimo nell'agosto 2019 e oggi siamo al dicembre 2020. Dopo tredici mesi avete stabilito che era necessario e urgente? Non ci siamo.

Stringiamo. Con Salvini si erano dimezzati; con il ministro Lamorgese si sono triplicati. Qualcuno, in Commissione, ha anche detto che non basta guardare solo i numeri, ma che c'è anche l'aspetto umanitario.

I numeri, cari colleghi, non valgono solo in termini di persone che arrivano. Purtroppo, c'è anche un onere economico da dover sostenere. Periodo del Governo Gentiloni: 2,2 miliardi. I fondi già erano stati dimezzati, rispetto ai 5 miliardi che spendeva Renzi.

Concludo con l'ultimo requisito, citato anche dal collega Balboni: la straordinarietà. Dev'esserci un caso straordinario.

ha il numero massimo di morti rispetto a tutta Europa. A livello mondiale, abbiamo superato il numero totale dei morti della seconda guerra mondiale.

aprire i porti, rendere più facile l'acquisizione del permesso di soggiorno e la conversione in un permesso di lavoro (che dev'essere dato anche a chi non ha lavoro).

Si è realizzato anche nei mesi precedenti, tranne che in un piccolo periodo, in cui ancora si applicava qualche legge. Se, però, l'incremento c'è stato, anche quando erano in vigore i decreti-legge Salvini, vuol dire che qualcuno non ha applicato la legge. A questo punto, se sia omissione di un atto d'ufficio oppure favoreggiamento di immigrazione clandestina, lo lascio decidere a voi, perché di questo è responsabile il Governo.

la dottrina prevalente ritiene che il sindacato sulla necessità e l'urgenza dell'atto sia di natura prettamente politica, anche se sono possibili esiti giurisdizionali. L'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 indica le ipotesi in cui non è possibile ricorrere al decreto-legge e non dobbiamo mai dimenticare che quello al nostro esame è stato emanato dal Presidente della Repubblica. Allora, se diamo per acquisiti questi fatti, e non può essere diversamente, dobbiamo svolgere un altro tipo di relazione e di osservazioni.

di chiarirne alcuni profili tramite una loro rimodulazione, che tenga conto dei principi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia. Questo è il punto del problema. I decreti Salvini confliggevano con i principi della nostra Costituzione e del diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 1, afferma che «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». della Dichiarazione universale dei diritti umani si afferma che il riconoscimento della dignità specifica e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della società umana è la base della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. I diritti umani rappresentano i diritti inalienabili che ogni uomo possiede; il diritto alla vita e ad un'esistenza dignitosa. Giovanni Maria Flick, che è stato anche evocato nel dibattito in Commissione da qualcuno di voi, Presidente emerito della Corte costituzionale, in un suo recente saggio breve, «Elogio della dignità», fa questa affermazione: «la dignità è premessa e condizione di eguaglianza e al tempo stesso di diversità; è espressione e frutto di solidarietà; è fondamento e limite

con straordinaria disinvoltura - direi con colpevole determinazione - l'avevano derubricata a fatto non essenziale. *Ex facto oritur ius*, come afferma un brocardo latino.

colleghi, signori del Governo, credo che sia arrivato il momento di sfatare una teoria che è stata più volte sostenuta in quest'Aula, secondo la quale in tempi di emergenza - in questo caso, sanitaria ogni provvedimento che esuli da quella strettamente pandemica debba essere bollato con un giudizio di inadeguatezza allo spirito dei tempi e alla necessità di fronteggiare l'aspetto principale, conseguente all'emergenza economica, dovuta alla diffusione della pandemia. Il Parlamento ha proseguito sempre la sua attività non si è mai fermato, non ha fatto un giorno di stop.

constatiamo nella quotidianità della nostra vita, pure in questo tempo di pandemia. Mi riferisco ai guasti causati dall'emanazione dei cosiddetti decreti Salvini.

o, meglio, non si può far finta di aver dimenticato i rilievi che sono stati immediatamente portati alla nostra attenzione dal Quirinale.

pubblicizzato di ridurre gli sbarchi; invece, com'è noto e come le statistiche ci dimostrano in modo inconfutabile, c'è stato un aumento di quegli sbarchi proprio durante la vigenza dei cosiddetti decreti sicurezza. Un'altra contestazione che dev'essere rispedita al mittente è quella degli irregolari, i quali - anche questa è stata un'emergenza - sono aumentati proprio dopo l'entrata in vigore - guarda caso - dei cosiddetti decreti sicurezza, decreti sicurezza, che avevano abolito la cosiddetta protezione umanitaria, aumentando in maniera esponenziale il numero delle persone che irregolarmente soggiornano nel nostro territorio. atto del fatto che l'urgenza esiste ed esisteva; questo provvedimento quindi interviene giusto per sanare quell'inefficienza e quelle ingiustizie.

ma, nello stesso tempo, era necessario, perché abbiamo da affrontare una stagione che purtroppo è ancora lunga e della quale ancora non conosciamo i tempi reali.

introdussero elementi che hanno perturbato la tranquillità e anche la sicurezza della comunicazione pubblica; mi riferisco, per esempio, alle notizie diffuse riguardo al contagio da parte degli irregolari. Questa è oggettivamente una menzogna, utilizzata per influenzare l'opinione pubblica e per creare e diffondere la narrazione di coloro che, in dispregio dei più elementari principi umanitari, hanno alimentato un quadro generale assolutamente fasullo. Da ultimo - come ricordavo in premessa - le modifiche che oggi apportiamo ai testi, di fatto rovesciandone il contenuto, non sono frutto di un capriccio o della volontà di affermare qualcosa di diverso rispetto alla maggioranza che ha voluto e sostenuto quei decreti.

hanno presentato da subito, che erano stati contestati nell'immediatezza da noi, che allora eravamo all'opposizione, e che sono tuttavia ancora presenti - aveva

ci si rende conto che può essere anche un semplice insegnante; è una norma quindi, anche quella, affetta da palesi dubbi di costituzionalità, perché non corrispondente a un principio di ragionevolezza. Per non parlare delle misure sproporzionate: un milione di euro di ammenda è evidentemente una sanzione che serve soltanto come *spot*,

Oltre alla lotta a quel virus invisibile, questo Parlamento, con la conversione del decreto-legge che speriamo di portare in porto nella giornata odierna, afferma principi di profonda attenzione intanto all'emergenza che viviamo, ma anche a tutti i problemi conseguenti all'emanazione e all'applicazione dei cosiddetti e riporta anche all'applicazione di un principio che la nostra Costituzione ci impone, quello del rispetto della persona umana,

dei requisiti di urgenza, ci pare davvero fuori luogo e soprattutto lontano dalle necessità di questo Paese nel momento gravissimo che stiamo vivendo e che dovrebbe richiamarci a un senso di più alta responsabilità.

non mi sto a dilungare sul problema che abbiamo oggi in quest'Aula, sulla questione dell'incostituzionalità sul fatto che il decreto-legge presuppone che ci siano i criteri di necessità e di urgenza. Questo l'ha già spiegato molto bene il collega Balboni. Vorrei farvi riflettere anche su un'altra questione che fino adesso è stata trascurata, cioè che il Presidente della Repubblica per firmare questo decreto-legge, come qualcuno di voi ricorderà, ci ha messo quindici

se il Presidente della Repubblica ci ha messo così tanto tempo a firmare questo decreto-legge. Credo che i criteri di necessità e urgenza,

scendere dalla luna e immergervi nel Paese reale! Questo dovreste fare. E invece no,

non è obbligatorio rimanere in Aula, mentre lo è consentire alla collega di svolgere il suo intervento. Anche la Presidenza fa fatica a seguire. Oltretutto, la mascherina non ci agevola. Prego, Presidente. Gli italiani, cari colleghi, non vi stanno chiedendo di abolire i confini; gli italiani non vi chiedono di aumentare il traffico nel Mediterraneo delle ONG e degli scafisti; gli italiani non vi chiedono di aumentare il fatturato delle cooperative che si occupano della gestione dei migranti. Non vi chiedono tutto questo e, soprattutto, non vi chiedono di aumentare i morti nel Mediterraneo, perché è questo che, con il vostro decreto, succederà.

Vi occupate di far diventare l'Italia il centro profughi d'Europa e di raccogliere tutte le miserie del mondo, senza dare le risposte agli italiani.

anziché rispondere ai tanti bisogni dei nostri connazionali, vi occupate dei clandestini, di incrementare il fatturato e di aumentare il traffico nel Mediterraneo. Vorrei concludere, signor se tante sarebbero le cose da dire. Sono fiduciosa negli italiani, che sapranno giudicare l'operato di questo Governo. Giudicheranno loro la distanza che avete con i bisogni delle persone. Giudicheranno loro il comportamento di questo Governo. Nella giornata di giovedì 18 dicembre,

non avete nemmeno ascoltato le parole della von der Leyen, quando ha detto che l'Italia deve assumersi la responsabilità

principale per l'emanazione di questo decreto, quindi la necessità e l'urgenza, fosse il ripristino dei principi costituzionali che erano stati violati sistematicamente, come vari interventi hanno dimostrato nel tempo, con i due decreti sicurezza, i cosiddetti decreti Salvini. Vi pare non necessario e non urgente ripristinare i principi costituzionali? Credo che sia questo il problema fondamentale. Non era un caso che il secondo decreto fosse accompagnato da una lettera del Presidente della Repubblica che diceva in modo molto chiaro quali erano gli elementi su cui intervenire e i profili di violazione costituzionale, a partire dall'articolo 10 della nostra Costituzione. Bastava solo e unicamente questo

ricordato il punto programmatico che ne parlava e siamo orgogliosi che questa maggioranza abbia tenuto fede all'attuazione di uno dei punti programmatici che le hanno dato vita.

c'è solo la violazione dei diritti e dei trattati internazionali, ma un danno vero. Quei decreti-legge, che pomposamente chiamavate decreti sicurezza, in realtà hanno prodotto solo e unicamente insicurezza.

conclusione, siamo tutti convinti che bisognerà intervenire nuovamente in modo complessivo, finalmente, su tutta la questione immigrazione e mettervi mano una volta per tutte

Signor Presidente, signor Vice Ministro, membri del Governo, colleghi e colleghe, ringrazio il mio Gruppo per avermi permesso di intervenire in questa discussione sulle pregiudiziali

lo stesso trattamento. Entrerò più nel merito. Il Presidente della Repubblica, come sapete - è stato citato più volte - ha mandato una lettera al Presidente del Consiglio nell'agosto 2019 parlando di una promulgazione con riserva, che non è una bocciatura, ma quasi. La promulgazione con riserva deriva da indicazioni precise che il Capo dello Stato dà in termini di necessità di proporzionalità tra sanzioni e comportamenti e di fondamentale conformità alle normative internazionali. Non è poco, è molto per un Paese come Italia che, nell'ambito degli accordi internazionali, è sempre stata in prima fila nel rispettarli e nel promuoverli. Inoltre, la Corte costituzionale rileva talune questioni sui decreti-legge sicurezza 1, sicurezza 2, Salvini - non so più come chiamarli in merito alla preclusione all'iscrizione anagrafica, che viene da sé, con un po' di logica e un minimo di ragionamento. È ovvio che se le persone non le riconosci, le stese saranno invisibili, e dove c'è l'invisibilità non potrà esserci niente di buono né per le persone invisibili né per tutti gli altri che vivono intorno. Questi sono i termini

L'umanità, la giustizia, l'importanza, la sacralità della vita non vengono mai meno e avranno per noi sempre rilievo di urgenza e di priorità.

di quest'Assemblea - metter fine alle speculazioni, perché, colleghi, laddove voi ci accusate di fare speculazione sulla vita delle persone che traghettiamo in mare (perché di questo ci accusate),

non faccia onore all'Assemblea e ai ruoli che rivestiamo stare così in basso e buttarsi nella mediocrità di queste accuse invertite che ci muoviamo in continuazione. Credo che il tema sia importante e che sia urgente riportare verità, che cioè non si debba parlare di insicurezza o di mancanza di sicurezza accostandola al migrante, al diverso, a una persona

Ogni Stato ha diritto di regolare i flussi migratori e di attuare politiche dettate dalle esigenze generali del bene comune, ma sempre assicurando il rispetto della dignità di ogni persona: il diritto della persona ad emigrare è iscritto tra i diritti umani fondamentali, con la facoltà di ciascuno di stabilirsi dove crede più opportuno per una migliore realizzazione

Questo ci dice che le migrazioni - ma lo sappiamo o comunque dovremmo saperlo - sono un fenomeno complesso, che è nella storia del mondo, dell'umanità, da migliaia di anni.

dire a noi stessi che il fenomeno delle migrazioni è complesso, e come tutti i fenomeni complessi richiede approfondimento, studio e quindi fatica,

Ho sentito delle cose veramente inenarrabili. È opportuno riportare la verità, ossia che dovremmo avere il coraggio di abbandonare le speculazioni e di dirci che la tutela dell'altro è importante e va fatta in modo serio, responsabile, costruttivo, e dovremmo sempre averla come priorità. Ho ancora un minuto. l'autrice del richiamo, che è assolutamente fuori luogo. Io sono convinta di quella che avevo già appurato e l'ho confermato riascoltando anche il mio intervento dell'agosto 2019, ossia il fatto che siamo diversi ontologicamente e per formazione. Per noi contano la vita, l'umanità, i diritti e la giustizia di ogni persona. Io potrei essere migrante un domani, come lei, Presidente, potrebbe esserlo dopodomani; ciascuno di noi, colleghi, in questo momento ha la fortuna di non dover migrare, ma non si sa mai cosa può succedere e quest'anno ce lo sta insegnando. Tutti noi potremmo trovarci un giorno a dover andare in un altro Paese per necessità o per scelta, perché pensiamo che lì potremmo avere una vita migliore. Questo è solo il primo passo - lo dico anche al mio partito - e ci aspetta molto di più per risolvere questo fenomeno. Non basta - mi rivolgo a lei, signor Vice ministro, e al Presidente, ma lei lo sa

di un impegno serio, costruttivo e responsabile. Noi ci siamo, ci dobbiamo essere. Per me e per il Partito Democratico questa resta una priorità urgente, e per questo motivo votiamo no alle questioni pregiudiziali.

del Governo, colleghi, spero che quello ad immigrare non sia un invito che dà anche una prospettiva futura al popolo italiano, perché vi dico che siete sulla strada giusta. *(Applausi)*. che questo provvedimento non passi, perché è lacunoso e non solo: è incostituzionale, mancano i presupposti di necessità e di urgenza. Soprattutto, vi voglio dire che sotto il profilo sostanziale, siccome si parlava di verità, mi permetterò di evidenziare alcuni elementi che spero faranno comprendere a quest'Assemblea le ragioni per le quali

State trasformando l'Italia in un grande campo profughi: è questa la verità. E voglio capire come mai, in un momento così delicato, nel quale stiamo affrontando notevoli problemi di carattere economico, problemi gravissimi e legati anche alla pandemia, come mai qualcuno crede che si possa pensare e immaginare che l'Italia possa essere recettiva. Di quanti? domanda, una domanda importante. Mi dovete dire qual è il limite dell'immigrazione in Italia.

10.000, 20.000, 50.000? Dateci un numero e poi, da sinistra, spiegate con le vostre fantasie e con la vostra immaginazione cosa dovremmo fare con quell'uno in più che arriva.

A chi ci ascolta diciamo che non c'è nemmeno bisogno dell'interpretazione dei politici; ci vuole lo psichiatra per capire come mai siete arrivati e vi siete spinti a tanto.

un meraviglioso giardino a cielo aperto, siamo un grande museo, siamo portatori di una civiltà straordinaria, quella greco-romana e giudaico-cristiana; siamo un punto di riferimento e - consentitemi di dire - di civilizzazione per le battaglie di libertà che abbiamo saputo portare e per il grande amore che abbiamo saputo anche donare alle nazioni, all'estero. Nessuno pensi, allora, che nel centrodestra vi sia o possa anche solamente albergare l'idea del razzismo o di qualcos'altro, che noi consideriamo un'infezione dello spirito. *(Applausi)*. Il razzismo è un'infezione dello spirito; lo voglio ribadire. Voglio anche dire, che raccontare a centinaia di migliaia di ragazzi che provengono dall'Africa che qui si può arrivare e trovare l'Eldorado, il paradiso terrestre è un atto che giudichiamo politicamente criminale. Non si può continuare su questa strada. Dovete rendervi conto della situazione nella quale viviamo. Siccome amiamo e vogliamo difendere questa Italia, vi diciamo che forse riuscirete anche a far passare questo provvedimento, ma noi, come

che questa abrogazione sarà - la saluteremo, se ci sarà - un momento molto importante e aggiungo che non capisco come mai, in un momento in cui il Governo ci viene a raccontare che siamo in zona rossa, che l'Italia rischia di trasformarsi in zona rossa, in cui non si potrà circolare da un paese all'altro,

in quella non dimenticata intervista ebbe a dire che si fanno più affari con l'immigrazione che non con la droga. È una vergogna!

è giusto accogliere chi scappa e chi viene perseguitato - sono principi che vogliamo continuare a difendere - dobbiamo anche dire con assoluta fermezza che chi viene in Italia per spacciare, combinare guai e finire nelle patrie galere non è giusto che permanga sul nostro territorio nazionale e deve essere assolutamente espulso. La nostra è una battaglia di fermezza in difesa dell'Italia e siccome il costo che stiamo sostenendo è un costo elevatissimo, vi invito a pensare e a ragionare sulla opportunità

perché immigrare non è un diritto, può essere un'aspirazione, per alcuni può essere una speranza, ma non è un diritto. Il diritto vero è quello di poter rimanere a casa propria, quindi con piani di investimento intelligenti operiamo in quella direzione. Ci sono Paesi, come ad esempio la Norvegia, che fanno grandi investimenti in Africa, ma hanno leggi estremamente severe nei confronti dell'immigrazione. Questa è una cosa che noi dovremmo cominciare a prendere in considerazione. Aggiungo che il nostro obiettivo, in Italia, dovrebbe essere - lo dico agli amici del centrodestra - di avere una legislazione sul modello di quella australiana,

Questo è il nostro obiettivo, un obiettivo assolutamente importante. Dovreste, per questa ragione, fare un semplicissimo raffronto di dimensioni. Potrei parlare di altri Paesi, ma mi limito all'Africa:

maggior parte giovani, che vogliono arrivare in Italia, hanno questa aspirazione di arrivare in Europa, ma noi sappiamo anche cosa accade purtroppo al nostro confine. Dobbiamo ricordarlo perché se non si contestualizzano le cose non si capisce qual è la situazione contestualizzare significa comprendere che se l'Austria ha chiuso i proprio i confini, se lo ha fatto la Francia, se lo hanno fatto tanti Paesi, noi ci troviamo in una condizione di estrema difficoltà.

e soprattutto, siccome abbiamo anche il timore e la preoccupazione che possano arrivare jihadisti o combattenti che tornano dal fronte siriano, avere in Italia (lo facciamo anche nell'interesse dell'Europa per la difesa dei nostri confini) confini) una legislazione sul modello di quella degli anni Settanta contro il terrorismo. Voglio dire di più, in conclusione. È necessario il blocco dell'immigrazione. Vogliamo arrivare ai respingimenti, vogliamo che chi arriva possa essere accolto dignitosamente, ma ma dobbiamo anche lanciare un appello a coloro che non amano l'Italia, ai tanti stranieri che hanno in odio la nostra lingua, la nostra religione, le nostre tradizioni, la nostra sicurezza, la nostra libertà. Ebbene, a costoro diciamo che l'Italia offre una grande libertà, un'altra grande opportunità, quella di tornare da dove sono venuti.

le richieste di improcedibilità o incostituzionalità del provvedimento. È inevitabile che su un provvedimento tanto controverso nasca una discussione politica anche in una fase squisitamente tecnica e questo dice quanto il Governo, con questo provvedimento, stia facendo anche carta straccia della nostra Costituzione. Premetto, però, che ho sentito alcuni interventi veramente bizzarri e mi riferisco innanzitutto a quello della senatrice Biti: Quando la senatrice Biti viene in Aula e parla di una legge che deve essere smontata per garantire i diritti umani, io chiedo: senatrice Biti, perché non era con me

Se fosse stato ancora ministro dell'interno Matteo Salvini, avreste chiamato i Caschi Blu per andare a Lampedusa! La vostra ipocrisia, però, è tale che definite come da disfare una legge che, quando è stata applicata, ha prodotto lo *stop* degli sbarchi dei clandestini in Italia e nascondete, invece, per comodo, la totale incapacità del Governo nella gestione dei flussi di migranti *(Applausi)* che porta, come ho visto a Lampedusa, ad avere i materassi messi all'aperto e la gente a dormire sotto l'acqua, o sotto il sole. Questo per voi è gestire l'immigrazione in maniera corretta? Questo per voi è rispettare i diritti umani? Questo per dire che questo il decreto-legge che voi avete portato in Senato e con cui volete smontare i decreti sicurezza è infarcito, dalla prima all'ultima lettera, di ipocrisia! rivolgo anche alla senatrice De Petris, per la quale provo rispetto, ma che mi fa molto specie quando viene a dire che abbiamo creato delle condizioni per cui gli immigrati, una volta giunti in Italia, sono diventati, in virtù delle nostre leggi, dei decreti sicurezza, invisibili. Bontà di dio, ma l'abbiamo vista la visibilità che voi intendete, quando abbiamo scoperto che l'attentatore di Nizza era sbarcato a Lampedusa, era andato a Bari, era tornato ad Alcamo e poi era andato a compiere l'attentato a Nizza! *(Applausi)*. Questa è la visibilità che voi volete dare agli immigrati che arrivano in Italia, con tutte le telecamere del mondo a darne cronaca, perché tutti hanno visto chi arriva a Lampedusa, tutti hanno visto la serietà di questo Paese nel gestire i confini d'Europa. Perché quello è il confine d'Europa. Questa è la visibilità che volete? Li avete fatti emergere: bravi! Complimenti! è un'altra ragione per non procedere all'approvazione del decreto in esame, che andrà a smontare i decreti sicurezza. E fa bene chi lo definisce decreto clandestini.

pensa che gli italiani non si accorgano di quanto sta facendo, perché presi, ovviamente, da ben altri problemi. Quindi, nottetempo, approvate un decreto-legge che smonta i decreti sicurezza. Come, però, ha correttamente ricordato il senatore Calderoli, esiste una Costituzione che prevede (o, adeguandoci alla situazione attuale, dovrei dire che prevederebbe) all'articolo 77 che «quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni». Presidente, io ribadisco, per la cronaca e per la conoscenza dell'Aula e anche di qualche senatore di maggioranza distratto, che il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto

proposte di modifica regolamenti, come regolamento Dublino III. Tali proposte prevedono, testualmente, di impedire gli spostamenti non autorizzati ai richiedenti all'interno dell'Unione europea stabilendo, fra l'altro, che questi ultimi dovranno presentare domanda nello Stato membro di primo arrivo

ancora non è scaduto il termine degli emendamenti e tuttora il Governo cerca in qualche modo di chiudere la porta all'opposizione, facendo già prefigurare l'imposizione della fiducia perché non volete che gli italiani sappiano che cosa state cambiando in questo decreto e volete farlo velocemente. Tuttavia, Presidente, ieri, durante l'audizione in Commissione ricordata, è emerso in maniera chiara che ci sono anche dei profondi vizi costituzionali. detto infatti dal professor Gaetano Carlizzi, si può sostenere senza alcun dubbio l'incostituzionalità per violazione degli articoli 3 e 117 della Costituzione e, ancora di più, dell'articolo 1, per la parte relativa che non prevede la retroattività e che dispone l'abolizione dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 12, comma 6. È evidente che quanto avete messo insieme non ha i requisiti di urgenza, non ha nemmeno i requisiti di omogeneità e non ha nemmeno la necessità di straordinarietà come ho appena argomentato. Emergono però ulteriormente anche delle incongruenze costituzionali relativamente agli articoli 3 e 117. Presidente, non si può procedere alla conversione in legge del decreto-legge. Quanto voi state facendo viola la Costituzione, i diritti dei cittadini regolarmente inseriti come stranieri in questo Paese, viola i diritti degli italiani. Non si può procedere.

sui temi che stiamo discutendo. Noi stiamo discutendo di immigrazione e siamo tutti lieti di aver appreso che in questi attimi è stata annunciata la liberazione dei pescatori siciliani, ingiustamente sequestrati in Libia. Il nostro Gruppo, ma anche gli altri, avevano chiesto nelle settimane passate una più incisiva iniziativa del Governo, che tardivamente pare sia giunta. Siccome però apprendiamo contestualmente che si sarebbero recati in Libia il Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari esteri, nell'esprimere grande gioia per questo evento, vorremmo anche capire dal Governo se la presenza del Presidente del Consiglio, quindi di un'autorità elevatissima, e del Ministro degli affari esteri, non abbia comportato accordi politici di varia natura, che sono connessi anche alle tematiche della sicurezza del Mediterraneo e dei flussi migratori. Vorremmo capire qualcosa di eventuali impegni assunti dall'Italia. Chiediamo chiarezza su questa vicenda, esprimendo gioia per la liberazione dei pescatori.

perché questo non può essere in alcun modo il risultato di una parte politica.

perché questo sarebbe intollerabile per un senso della misura che tutti noi siamo tenuti ad osservare.

è una notizia su cui l'Assemblea non può che esprimersi con un rallegramento e con la sottolineatura del fatto che si tratta di un risultato per il nostro Paese e per l'impegno istituzionale di tutto il Parlamento.

di Mazara del Vallo sono stati liberati e speriamo che presto possano rientrare, grazie all'impegno del Presidente del Consiglio e del Ministro degli esteri. Io credo che questo sia un avvenimento che ci deve vedere gioire, a prescindere dalla parte politica che ognuno di noi rappresenta. Per cui ringrazio il Governo per l'azione svolta e ringrazio anche il Parlamento, che ricordo che in queste settimane, nei giorni di vera e propria detenzione, ha svolto un ruolo di pungolo costante, con interventi nelle sedute di *question time*, con interrogazioni e con interventi in tutti i provvedimenti che sono stati approvati in quest'Aula. Tutte le forze politiche hanno rappresentato il loro sostegno al Governo affinché potesse svolgere questa azione celermente. Grazie a tutti i parlamentari di quest'Aula e un grande abbraccio ai familiari, che hanno sofferto tantissimo.

Signor Presidente, ovviamente a nome di Fratelli d'Italia siamo felici, perché sembrerebbe che questa detenzione, durata centosei giorni, oggi finisca. Purtroppo l'Assemblea non può oggi non ricordare l'umiliazione che questo Governo di inetti ha inflitto alla nostra Nazione.

pescatori nell'arco di pochi giorni. *(Applausi)*. Ricordiamo che un'analoga situazione è accaduta alla Turchia di Erdoğan, che ci ha messo cinque giorni a liberare i suoi pescatori.

e il nostro Ministro degli affari esteri volano a Bengasi e mi auguro, per il bene della nostra Nazione, che nessuno poi voglia vantarsi di aver riportato a casa, con cento giorni di ritardo, i nostri pescatori. Per concludere la figuraccia internazionale che l'Italia ha fatto per questo Governo di inetti, ricordiamo le dichiarazioni del Governo che ha più volte detto che la nostra *intelligence* era al lavoro. L'*intelligence* si adopera quando c'è un sequestro, non quando dei pescatori sono detenuti in un carcere di un Paese noto. Se i nostri Servizi segreti devono scoprire dove sono i pescatori, non siamo messi bene.

Questa gente qui che non è riuscita in cento e otto giorni a farsi consegnare dei pescatori da uno Stato libico vorrebbe intimidire me; dai, facciamo i seri un attimo. Con tutto il ritardo e tutta la vergogna ci auguriamo che il Ministro degli affari esteri e il *Premier* non si rivendano questa vergogna come una vittoria. una nuova finestra"). Presidente La Russa, ci sono altri senatori che sono iscritti a parlare prima di lei. Il suo Gruppo è già intervenuto, quindi aspetterà anche lei un momento e poi valuteremo, essendo già intervenuto un rappresentante

Mi rendo conto che l'Italia è un Paese particolare, un Paese strano, ma oggi oggettivamente mi sembra paradossale che un senatore di un Gruppo parlamentare che si chiama Fratelli d'Italia si comporti in questa maniera nel giorno in cui tornano a casa i nostri pescatori. Si comporta in questa maniera, dando addosso all'operato del Presidente del Consiglio, del Ministro degli affari esteri, di tutto il Governo e di tutto il Parlamento, quando dovremmo ricordare che non è possibile che, nei casi in cui il nostro Governo si comporta finalmente in maniera autorevole, non solo nel Mediterraneo ma nel contesto internazionale, è merito di qualcuno e quando invece ci sono situazioni difficili è sempre colpa del Governo. Da più parti viene chiesto un atteggiamento più assertivo dell'Italia, ma l'Italia ha una Costituzione e questo Parlamento la segue e la rispetta e la rispetta come fa anche il Governo. La questione dei nostri pescatori ha dimostrato che l'atteggiamento pacato e cauto, ma in continuo contatto con la nostra *intelligence* porta risultati per un Paese che non può e non deve assumere iniziative di guerra per riportare a casa le proprie persone. *(Applausi)*. Abbiamo una Costituzione e la dobbiamo rispettare, ma non siamo un Paese che si può permettere atteggiamenti del genere nel Parlamento nazionale. Abbiate la decenza di rispettare quello che è successo oggi, e ringrazio i colleghi che lo hanno Grazie a tutti

Quella di oggi deve essere una giornata di festa per tutti, se così sarà, senza distinzioni politiche e partitiche. Sottolineo una preoccupazione che spero si riveli infondata, visto che sono stato Ministro dell'interno. L'operazione che sta andando a compimento (ma in queste operazioni servono estreme cautela e riservatezza)

la mia seppur breve esperienza al Governo mi insegna che queste operazioni si annunciano a pescatori a pescatori rientrati in Italia. Non vorrei - e Dio non voglia - per rispetto delle famiglie che sono non solo italiane, ma senegalesi, tunisine e bengalesi (perché sulle nostre navi l'integrazione è realtà, non chiacchiere), che - e spero di essere smentito - un'operazione a cui lavoravano da settimane i nostri Servizi di sicurezza...

che decide cosa deve dire o non dire il Presidente del Consiglio (ogni riferimento a Casalino è puramente casuale e voluto)

Visto che l'operazione, se andrà a buon fine (e lo spero per i familiari di questi lavoratori), sarà grazie ai nostri Servizi segreti (come si sarebbe detto una volta), è squallido, vergognoso e irrispettoso che perfino sui giornali si legga che oggetto della verifica del rimpasto di maggioranza sono le nomine ai vertici dei Servizi segreti. *(Applausi)*. È una cosa indegna di una democrazia sviluppata. Viva i nostri pescatori e chi lavora in silenzio senza danneggiare gli sforzi altrui!

di questi uomini e per la risoluzione di un problema internazionale molto, molto rilevante. Il merito è del Governo, è dell'*intelligence*, è del Parlamento e del Paese intero che è stato vicino a queste persone e a queste famiglie. *(Applausi)*. fare confusione in un giorno come questo è semplicemente sbagliato. *(Applausi)*.

ci sia stata una cagnara incredibile senza che nessuno venisse richiamato all'ordine. Gli altri hanno potuto parlare tranquillamente.

Signor Presidente, mi duole rappresentare ancora una volta in quest'Aula il disappunto mio e del mio schieramento in relazione a dinamiche ricorrenti che vedono Gruppi di opposizione rappresentare questioni pregiudiziali dal contenuto - consentitemi di dirlo - vuoto (in seguito argomenterò) e prive di particolare significato. Sia ben chiaro - ci tengo a precisarlo - che questo disappunto non è una critica al dibattito parlamentare parlamentare ma allo svilimento di strumenti che potrebbero essere utilizzati per innalzare il livello del dibattito e non, ancora una volta, come accade oggi, per asservirli a intendimenti propagandistici e ce ne siamo accorti. Avevo qualche dubbio ad intervenire in discussione sulle pregiudiziali. Pensavo di essere in discussione generale visto che gli argomenti trattati non riguardavano assolutamente l'oggetto della discussione. Millantare l'incostituzionalità di un decreto adottato per superare i profili di costituzionalità sollevati dal Presidente della Repubblica è sinonimo di mancanza di serietà del dibattito parlamentare. Dichiarare nero su bianco la disomogeneità di un provvedimento i cui contenuti sono similari a quelli dei decreti precedentemente adottati da chi ora siede sugli scranni dell'opposizione non favorisce certo il recupero della centralità del Parlamento in un sistema istituzionale in cui l'organo titolare del potere legislativo chiede a gran voce di recuperare un peso specifico che possa influire nelle dinamiche politiche contingenti. Un dibattito parlamentare serio non metterebbe in dubbio, con questioni pregiudiziali, un provvedimento nato proprio per superare i problemi di costituzionalità prodotti dalla decretazione precedente e fatti valere

dell'8 agosto 2019, che ha richiamato il principio generale della proporzionalità tra sanzioni e comportamenti, definito necessario nella sentenza n. 112 del 2019 della Corte costituzionale, e la necessaria conformità alla normativa internazionale, a partire dalla Convenzione di Montego Bay, tanto citata nelle Ancora, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2020, ci dice testualmente che, a dispetto del dichiarato obiettivo dell'intervento normativo di aumentare il livello di sicurezza pubblica, la norma in esame, impedendo l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, finisce con il limitare la capacità di controllo e il monitoraggio dell'autorità pubblica sulla popolazione effettivamente residente sul territorio. garantire il tempestivo ripristino del rispetto del diritto di accoglienza e ripristinare i principi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia, ponendo rimedio a tutti gli aspetti funzionali, che causano difficoltà applicative, in un momento già di per sé complicato, che non fanno altro che generare ulteriore *caos*, rendendo difficile la gestione dei nuovi flussi. Per di più, il decreto in esame è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento, nel quale i profili di costituzionalità, inclusi il riparto delle competenze fra Stato e Regioni, così come la necessità, l'urgenza e l'omogeneità contenutistica, sono già stati attentamente vagliati. Si deduce quindi che non sussistono problemi di legittimità costituzionale e che, come ho detto prima, si tende proprio a superarli. Anzi, la nostra Costituzione ha ha al centro la dignità della persona e, per quanto riguarda i diritti fondamentali, pone sullo stesso identico piano il cittadino e lo straniero, rafforzando il concetto dell'articolo 10. Prendiamo atto in quest'Aula, non è urgente onorare la Costituzione. Cari colleghi, il mio invito è quello di tornare a fornire contributi concreti e contenuti solidi e migliorativi dell'operato della maggioranza di questo Paese, che è da sempre aperta al confronto e al dialogo costruttivo con le opposizioni, ai fini del recepimento di idee proficue e per il bene di tutti. *(Applausi)*.

ho personalmente visto il senatore Vitali votare per due. *(Proteste).* Capisco che la senatrice Papatheu stia sotto, però un senatore non può essere delegato da un altro senatore. Quindi, la prego

ai fini della diaria, i senatori che inseriscono soltanto la tessera non si vedono decurtata quella somma che andrebbe invece

abbiamo contezza delle presenze in Aula e dell'allineamento, quindi se ci sono voti per altri viene segnalato anche dai segretari e la Presidenza interviene immediatamente.

recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131*-bis*. 391*-bis*, 391*-ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

Signor Presidente, le chiederei un'ora di tempo per poter riunire le Commissioni. Abbiamo svolto i nostri lavori nella giornata di ieri fino a tarda

faccio presente che, come ha già riferito il presidente Parrini, siamo convocati

Mi pare che sia stata data contezza esauriente dello stato dei lavori delle Commissioni riunite. Tra l'altro, c'è una coincidenza anche sull'esigenza dei tempi di sanificazione dell'Aula,

2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131*-bis*, 391*-bis*, 391*-ter* e 588 del codice penale, nonché misure in misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private

nello spirito di collaborazione che porterà all'approvazione del provvedimento nella giornata odierna, accettiamo la richiesta *(M5S)*. Signor Presidente, anche noi riteniamo che un'ora sia un arco temporale adeguato per procedere nel modo più sereno possibile. Va bene anche per il MoVimento 5 Stelle.

La seduta è sospesa.

oggi siamo arrivati in fondo ed è un successo che, vorrei dirlo in premessa, secondo me non va ascritto ad un partito soltanto; e non è la rivalsa, come pure qualcuno

È anche un successo per tutta quella parte di Paese che guarda, con fiducia e con speranza, a una politica che vuole governare i problemi più grandi e difficili del presente, senza usarli mai per scopi partigiani né per affermare forza o proprio consenso. Oggi, con questo provvedimento, proviamo a chiudere una pagina aperta due anni fa sull'onda di una sbandierata emergenza e soprattutto, secondo me e secondo noi, sull'errata equazione immigrazione uguale insicurezza. Una pagina che, però, in questi due anni si è rivelata nei fatti sostanzialmente inefficace. Con questo provvedimento che, certo, sì, lo voglio dire con chiarezza, rivendica una scala di valori e una visione dei temi trattati differenti e nettamente alternativa, si apre una pagina diversa, ispirata a valori di solidarietà che uno Stato di diritto e democratico, come il nostro, dovrebbe avere sempre incisi nel proprio DNA. Questo decreto è un primo passo e non sempre i primi passi sono agevoli e semplici. La discussione è stata molto lunga alla Camera ed anche qui, seppure l'esame poteva apparire una semplice formalità, così non è stato. Detto questo, è evidente che il provvedimento rappresenta di certo un punto qualificante per l'azione del Governo. Il motivo è oggi esattamente lo stesso del 2019, quando questa compagine di Governo è nata proprio sull'idea che i cosiddetti decreti sicurezza Salvini andassero modificati, proprio perché nei fatti stavano ottenendo esattamente l'obiettivo contrario a quelli che si dicevano essere gli obiettivi invece dichiarati; non il controllo dei flussi, ma semplicemente più insicurezza e più illegalità per i cittadini e per i migranti. Come tutti sappiamo e come è stato anche ricordato, pesava, pesa e peserà sempre su di noi il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica,

internazionali. È stata richiamata anche stamattina la pronuncia della Corte costituzionale che aveva dichiarato illegittima la norma che esclude i richiedenti asilo dall'iscrizione anagrafica. Una norma

che quei due decreti nei fatti hanno prodotto: un esercito di persone in carne ed ossa emarginate, sbattute fuori dai percorsi di integrazione, depotenziate e gettate scientemente in zone d'ombra pericolose, costrette a vivere in un limbo e nella precarietà. Quei decreti insomma, al di là delle intenzioni dichiarate, hanno portato il nostro Paese fuori dalle regole condivise del diritto internazionale, allontanandolo dalla posizione che negli anni precedenti l'Italia aveva sostenuto anche in Europa per un impegno più coraggioso sulla gestione di un fenomeno tanto complesso e portandolo invece drammaticamente più vicino a Paesi, che rivendicavano il disprezzo delle regole basilari della nostra democrazia. In questo contesto mi sia consentito, anche in qualità di relatrice, un semplice inciso: mi chiedo come si fa in questa Aula, ma anche nel Paese, ad essere, da un lato, i più convinti sostenitori

soltanto da chi non persegue la totale chiusura dei confini nazionali, da chi accetta la fatica di governare il processo migratorio e non cerca invano di costruire muri di carta. Dico che oggi con questo provvedimento noi scegliamo di mettere fine al tempo delle semplificazioni. È arrivato il momento di lasciarsi alle spalle banalità come difensori dei confini, da un lato, e responsabili dell'invasione, dall'altro. È una retorica che ha avuto effetti disastrosi sulla percezione diffusa delle migrazioni: globale ed enorme del nostro tempo che riguarda tutti i Paesi. Non lo dico io. Sono i numeri - se solo si avesse la pazienza e l'umiltà di leggerli - a dire che l'andamento dei flussi nel Mediterraneo purtroppo è condizionato da fattori che solo in piccola parte hanno a che fare con le legislazioni nazionali. Penso allora che su un tema di questa portata l'obbligo per tutti noi sia rifuggire da banalità. Credo che ci sia anche però un nostro obbligo a rivendicare la responsabilità della politica di difendere una chiara gerarchia di valori. il primo posto vada al diritto alla vita, all'obbligo di rispondere al grido di aiuto soprattutto di chi viene e di chi è disperso in mare, di chi fugge da situazioni di difficoltà inaccettabili, che mettono a rischio la propria vita. Ecco perché è inaccettabile l'atteggiamento di chi trasforma le Organizzazioni non governative, che prestano attività di soccorso in mare, nei responsabili di tragedie, come se le ONG fossero i protagonisti al soldo di non so quale finanziatore. Non è accettabile perché è un dato falso, come dimostrano anche i procedimenti giudiziari avviati Grazie a tutti quei rischi per la sicurezza derivanti dalla privazione di qualsiasi identità, qualsiasi diritto e qualsiasi dovere. Lo si fa modificando la procedura di esame prioritario accelerato delle domande di riconoscimento della protezione internazionale, che significa di fatto subire una contrazione significativa del diritto di difesa. Aggiungo anche che aver escluso le vittime di tratta da questa procedura accelerata significa dare una tutela minima a donne che vivono già in una condizione davvero di estrema disperazione. E allora ripariamo allo strappo consumato sul piano dell'accoglienza prevedendo che tutta una serie di permessi di soggiorno, tra cui quelli per gravi patologie, consentano poi di lavorare. Viene esteso il divieto di rimpatrio, con un'attenzione specifica ai soggetti più vulnerabili, anche in base all'orientamento sessuale. Si prevede inoltre un permesso speciale nei confronti di colui quale vale il divieto di espulsione ed è senza protezione internazionale; è il modo per evitare che lo straniero privo di forme di protezione codificate resti in una zona grigia senza un titolo legittimo di soggiorno. Si riduce il tempo per l'ottenimento della cittadinanza e si elimina il termine attuale del decreto flussi. È inserito l'obbligo per i prefetti di sentire i sindaci prima di aprire nuovi centri di accoglienza e si continua nell'azione di tutela e integrazione dei minori stranieri non accompagnati. Voglio dire che sono tutte norme giustificate dall'idea, che mi pare abbastanza ragionevole, che è meglio conoscere piuttosto che chiudere gli occhi, è meglio riconoscere una posizione piuttosto che gettare in una zona d'ombra, è meglio integrare piuttosto che escludere ed emarginare. Questa è la differenza più visibile rispetto al recente passato. Anziché provare inutilmente a chiudere il nostro Paese di fronte a un fenomeno epocale, noi proviamo con questo provvedimento a rimetterlo nelle condizioni migliori per gestire un fenomeno complesso, attraverso un sistema di accoglienza diffusa e inclusione sociale, evitando concentrazioni di persone e di interessi, puntando invece sulla distribuzione sul territorio di richiedenti asilo e beneficiari di protezione. Anziché rendere invisibili le persone che arrivano dobbiamo favorire percorsi di formazione e integrazione e incentivare che si partecipi ad essi con impegno. Ho detto ovviamente che questo è solo un primo passo; altri ne dovremo fare. ho detto poi all'inizio, questo non è il successo di una parte, anche se una parte ovviamente ha condotto con più coerenza, determinazione e convinzione questa battaglia. Oggi con questo provvedimento si afferma l'idea di un Paese che non crede che distinguendo gli ultimi da altri ultimi, come pure ho sentito nella discussione in questi ultimi giorni in Commissione, ne proteggiamo meglio alcuni, che non è mettendo ultimi contro altri ultimi che si mette in sicurezza un sistema Paese oppure semplicemente le certezze di chi è più fortunato o garantito. Oggi con questo provvedimento, a mio avviso, a vincere non sono solo valori di umanità, solidarietà, rispetto e dignità per tutti, ma è anche l'idea che solo attraverso tutele, opportunità e diritti sacrosanti riconosciuti a tutti, solo attraverso un'effettiva riduzione di divari, disuguaglianze e marginalità sociali e quindi solo attraverso integrazione, partecipazione e riconoscimento a tutti di pari dignità si costruiscono sistemi e comunità più forti, più competitive, più sane, ma soprattutto comunità più sicure per tutti.

Per quanto riguarda la parte relativa alla Commissione giustizia, il testo di legge che oggi siamo chiamati ad approvare, all'articolo 6, consente l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita anche con riguardo ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza. L'articolo prevede che, per i medesimi delitti indicati nel comma 7-*bis*, si proceda sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. L'articolo 7, intervenendo sull'articolo 131-*bis* del codice penale, limita il campo di applicazione della preclusione all'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto nelle ipotesi di resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. La modifica è volta a circoscrivere la preclusione ai reati commessi non più nei confronti di un pubblico ufficiale, ma nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni. Contestualmente, la disposizione preclude sempre l'applicazione della tenuità del fatto alle ipotesi di oltraggio a magistrato in udienza. L'articolo 8 invece interviene sull'articolo 391-*bis* del codice penale allo scopo di inasprire il regime sanzionatorio per chiunque agevoli nelle comunicazioni con l'esterno il detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario. La pena base diventa la reclusione da due a sei anni in luogo della reclusione da uno a quattro. La pena per la fattispecie aggravata diventa la reclusione da tre a sette anni in luogo della reclusione da due a cinque anni. È inoltre estesa l'applicabilità delle medesime pene anche al detenuto che, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis*, comunica con altri in violazione delle prescrizioni imposte. L'articolo 9 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 391-*ter* per punire con la reclusione da uno a quattro anni chiunque mette a disposizione di un detenuto un apparecchio telefonico. La fattispecie si applica anche al detenuto che usufruisce del telefono e specifiche aggravanti sono invece previste quando il reato è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio e anche da un avvocato. L'articolo 10 modifica l'articolo 588 del codice penale che punisce il reato di rissa, inasprendone le pene tanto per la fattispecie base, consistente nella partecipazione a una rissa, quanto per quella aggravata, che si applica quando, in conseguenza della rissa, taluno rimane ucciso o riporti lesioni gravi; si tratta della cosiddetta norma Willy, in memoria del povero Willy Monteiro Duarte di Colleferro, ucciso a pugni e calci in una rissa. L'articolo 11, modificando gli articoli 13 e 13-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2017, amplia l'ambito di applicazione delle misure del divieto di accesso ai locali pubblici o ai locali di pubblico intrattenimento (il cosiddetto Daspo) che possono essere disposte dal questore o autorità di pubblica sicurezza nei confronti di coloro che sono stati denunciati per specifici reati e inasprisce le sanzioni in caso di violazione dei suddetti divieti. L'articolo 12 implementa gli interventi per il contrasto del reato di traffico di stupefacenti, commesso attraverso l'utilizzo della rete Internet, prevedendo per i *provider* l'obbligo di introdurre strumenti di filtraggio dei siti *web* segnalati come strumento per la commissione dei suddetti reati e conseguentemente sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi. L'articolo 13 interviene infine sulla disciplina del Garante nazionale delle persone private della libertà personale, attribuendogli funzioni nell'ambito della prevenzione della tortura. Inoltre, si consente al Garante di delegare l'esercizio di alcune circoscritte funzioni ai garanti territoriali, quando particolari circostanze lo richiedano, per una durata massima di sei mesi. Infine, il mandato dell'attuale Garante è prorogato di due anni. Concludo, Presidente, ricordando a tutti che salvare vite umane è un nostro dovere giuridico, ma anche morale, e che l'accoglienza e integrazione dei migranti nel nostro Paese è un'azione che nobilita il popolo italiano, noto per il suo spirito altruista e solidale. Gli interessi e i diritti dei cittadini sono comunque sempre tutelati, come ha dimostrato questo Governo in quest'anno di emergenza sanitaria, a trecentosessanta gradi, con tutti i numerosi decreti emanati fino ad oggi. Il livello culturale e civile di un popolo si misura anche in base al livello di integrazione culturale che lo stesso offre.

il provvedimento che siamo chiamati a convertire non merita l'urgenza con cui si sta affrontando questa discussione. La nostra Costituzione prevede, all'articolo 77, comma 2, che il Governo possa adottare, in casi straordinari di necessità e urgenza, provvedimenti aventi forza di legge e la Corte costituzionale ha più volte ribadito l'illegittimità del decreto-legge che nel suo contenuto non rispetti il criterio di omogeneità, vincolo e presupposto essenziale per l'esercizio della decretazione di urgenza.

Sono altre le urgenze per il nostro Paese, che sta vivendo un momento particolarmente difficile, gravato dall'emergenza sanitaria e dalla crisi economica legata alla diffusione del Covid-19, e che avrebbe bisogno di interventi seri e concreti a sostegno dei cittadini e delle tante imprese che stanno soffrendo incredibilmente. I cittadini non hanno bisogno di disposizioni volte alla riapertura dei porti e dei confini; non hanno bisogno di un decreto clandestini. Il decreto-legge all'esame si rivela quindi del tutto estraneo rispetto alla realtà e alle reali necessità del Paese e addirittura irrispettoso nei confronti dei cittadini italiani. non è necessario, anche a fronte delle osservazioni del Presidente della Repubblica contenute nella lettera inviata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione. In tale lettera i rilievi relativamente alla materia dell'immigrazione riguardavano solo l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di violazione del divieto di ingresso nelle acque territoriali. Le azioni davvero necessarie in tema di immigrazione sarebbero dovute essere quelle volte a una riduzione del numero di clandestini che si riversa nel nostro Paese. Solo questo poteva essere un segnale chiaro e inequivocabile di presa di posizione da parte dell'Italia per dire per dire no alla tratta di esseri umani e per riacquistare credibilità agli occhi dell'Europa, agendo con politiche migratorie controllate volte a impedire che persone arrivate illegalmente sul nostro territorio vadano ad alimentare il fenomeno della delinquenza o addirittura del terrorismo, come ci hanno dimostrato i recenti fatti accaduti a Nizza poco più di un mese fa.

e ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Superfluo aggiungere altro. Il precedente Governo era riuscito finalmente a contenere i flussi migratori illegali e questo è un dato certo. Ciò che spesso si sottovaluta - o, meglio, si strumentalizza - è la conseguenza che da ciò deriva: diminuire il numero delle persone che arrivano illegalmente nel nostro Paese significa diminuire il numero delle persone che regolarmente muoiono cercando di affrontare un viaggio ai limiti della sopportazione umana. Un serio piano politico in materia di immigrazione non può basarsi su un'accoglienza indiscriminata, perché in questo modo non si riesce a garantire il giusto sostegno a quei migranti che avrebbero il diritto di essere accolti perché perseguitati o scappati da guerre civili. I decreti sicurezza che questo provvedimento stravolge tendevano a un'accoglienza mirata e ad avviare un processo di integrazione che prevede diritti, ma anche doveri per chi arriva nel nostro Paese e soprattutto per chi ha diritto di essere accolto. Il precedente Ministro dell'interno si è battuto affinché fossero organizzati i corridoi umanitari e che non fossero le ONG a gestirli perché non è loro compito. Deve essere lo Stato a farsene carico e questo presuppone azioni serie, mirate e ordinate e un'immigrazione governata da regole chiare anche per chi arriva nel nostro Paese. Le misure che leggiamo invece in questo provvedimento sembrano mosse da una finta volontà di integrare che è lontana dal potersi definire accoglienza. Entrando nel merito del provvedimento, all'articolo 1 si è modificata la disciplina del decreto flussi, introdotta nel 1998 dalla cosiddetta legge Turco-Napolitano, con la soppressione del termine previsto per la programmazione triennale da parte del Governo sulla base delle esigenze del mercato del lavoro e del limite delle quote stabilite nel decreto emanato nell'anno precedente. decreto sicurezza aveva sostituito il permesso di soggiorno per motivi umanitari (un *unicum* nel panorama europeo che si prestava, in assenza di una puntuale normazione, a un uso per questo a un uso per questo arbitrario) con permessi di soggiorno speciali, puntualmente disciplinati (condizioni di salute di eccezionale gravità, situazioni contingenti di calamità nei Paesi di origine, atti di particolare valore civile). Il provvedimento in esame amplia i casi in cui può essere concesso un permesso di soggiorno per calamità - una delle tipologie introdotte dal primo decreto sicurezza in sostituzione della protezione umanitaria - da contingenti ed eccezionali a solo gravi ed elimina il termine massimo di sei mesi per il rinnovo, che quindi potrà non avere limiti. Su questo punto si potrebbe aprire un dibattito. I permessi per calamità, già previsti dal decreto Salvini, erano legati a casi eccezionali e per calamità eccezionali e contingenti, come ad esempio il terremoto di Haiti o lo tsunami in Indonesia.

Rimane pertanto da stabilire quali siano le gravi calamità cui si allude, perché potrebbe verosimilmente trattarsi anche di siccità, di caldo eccessivo o di altre condizioni ambientali caratteristiche di alcuni Paesi. In questo modo potremo avere una nuova fattispecie di migranti: i migranti climatici. C'è da pensare attentamente a questo concetto. L'80 per cento dell'Africa subsahariana ha problemi di siccità, ma non sembra attuabile la migrazione dei 2,5 miliardi di persone che vivono in zone disagiate del nostro pianeta verso le nostre coste, né tantomeno una loro successiva regolarizzazione. L'articolo 1 consente, inoltre, lo svolgimento di attività lavorativa in caso di permesso di soggiorno per cure mediche, in modo irragionevole, considerata la specificità di tale permesso di soggiorno e il fatto che il titolare dovrebbe essere in condizioni di salute gravi. Si prevede poi la conversione automatica in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di una serie di permessi precedentemente esclusi (protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto di cittadinanza, attività sportiva, lavoro artistico, motivi religiosi, assistenza minori), senza alcun limite e di fatto sradicando tutta la programmazione dei flussi migratori. Questo è un punto che è importante sottolineare. Il permesso di lavoro viene dato a chi ha il permesso per residenza elettiva, il permesso per residenza elettiva, oggi concesso a coloro che hanno una pensione italiana, che dimostrano di essere autosufficienti e che non hanno bisogno di lavorare. Sembra paradossale, ma con questo provvedimento si vuole accordare un permesso di lavoro a qualcuno che deve dimostrare che non ha bisogno di lavorare. Siamo arrivati all'assurdo. *(Applausi)*. Lo stesso vale per il permesso per motivi religiosi che, per definizione, è rilasciato per soggiorni brevi. Anche questo può essere trasformato in permesso di lavoro. Il comma 1 reintroduce la possibilità del rilascio di permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, anche senza il parere del Ministro del lavoro - già abrogato dal primo decreto sicurezza - che quindi avverrà in automatico e senza alcun controllo. Inoltre, è stato soppresso il limite temporale, nonché le quote stabilite per il decreto flussi annuale, mentre si è disposto un ulteriore ampliamento dei motivi di non respingimento ed espulsione fino a ricomprendere l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Con il fine di incrementare il fenomeno migratorio nel nostro Paese e di agevolare le organizzazioni non governative, il provvedimento interviene eliminando dal testo unico sull'immigrazione la facoltà del Ministero dell'interno di poter limitare o vietare il transito di navi in mare territoriale,

Nella pratica il Governo vuole dare una legittimazione all'opera di traghettamento nel Mediterraneo svolta regolarmente dalle ONG. Il comma 2 inserisce nel codice della navigazione la facoltà di limitare e vietare solo la sosta e il transito in mare territoriale

da 10.000 a 50.000 euro, anziché da 150.000 a un milione di euro, come previsto dal decreto sicurezza bis: direi un bel regalo a Carola Rackete e ai suoi soci. Nel decreto Salvini si vietavano dunque l'ingresso e la sosta all'interno delle acque territoriali. In questo provvedimento non è più presente la parola «ingresso», per cui sono vietati solo la sosta nelle acque territoriali o il transito, mentre è consentito quindi evidente che il Ministro dell'interno, che resta comunque autorità di pubblica sicurezza, non può più vietare l'ingresso nelle acque territoriali. L'articolo 2 interviene sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Il comma 1 riformula le ipotesi di esame prioritario delle domande di asilo, ossia con precedenza, dandone competenza al presidente di commissione, assieme all'individuazione dei casi di procedura accelerata. A seguito della novella, per i casi di richiedente sottoposto a trattamento nei CPR o in un *hotspot*, perché richiedente asilo che non è possibile identificare, e di richiedenti provenienti da Paesi di origine sicura, viene eliminata la possibilità di procedere ad un esame prioritario della domanda. dispone altresì che, in caso di domanda reiterata, in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, si demanda la valutazione di ammissibilità al presidente della commissione, anziché operare automaticamente, ossia essere considerata inammissibile già dal momento della sua presentazione, come strumentale ad evitare il rimpatrio. La norma allunga la durata del permesso di soggiorno speciale, ossia la protezione umanitaria, da un anno a due anni, esattamente com'era prima del primo decreto sicurezza. A tale riguardo, prima della riforma di tale decreto sicurezza, su circa 40.000 tutele umanitarie riconosciute dalla commissione territoriale, dal 2015 al 2018, poco più di 3.200 sono state le conversioni in permesso di lavoro e circa 250 i ricongiungimenti familiari. La gran parte degli immigrati è rimasta in Italia inoperosa, senza concrete prospettive di stabilizzazione e di inclusione sociale, con il forte rischio di cadere in percorsi di illegalità. I titolari di protezione internazionale palesemente fondata, nel giro di pochi giorni vedevano avviato il processo di integrazione, perché le commissioni prefettizie autorizzavano il permesso di restare nel nostro Paese. Per tutti gli altri, che non avevano diritto di rimanere, come ad esempio tutti i migranti economici (attualmente un terzo degli sbarchi è composto da cittadini tunisini) era previsto un esame preliminare e la permanenza obbligatoria nei CPR, fino all'espulsione. Il nuovo testo elimina la formula «palesemente fondata» e apre a tutte le possibili interpretazioni della formula «ad una prima valutazione verosimilmente fondata». Una norma così aleatoria appare volutamente priva di sostanza, così come la formula utilizzata per autorizzare a rimanere sul nostro territorio

Concludo, signor Presidente. Inoltre si è preferito eliminare il riferimento esplicito alla tortura e ai trattamenti inumani o degradanti, per lasciare spazio al giudizio soggettivo di chi si trova a prendere la decisione. la protezione umanitaria, eliminata con i decreti Salvini, era un *unicum* in Europa, che non esisteva e non esiste in alcun altro Paese europeo. Solo in Germania c'è un istituto simile, ma per casi specifici, e il ministro Salvini aveva lavorato nella stessa direzione, per casi specifici.

quale tipo di obiettivo vi ponete, cioè quale modello avete davanti agli occhi e cosa volete fare del nostro Paese per i prossimi Questa è la domanda, perché con un decreto-legge del genere è chiaro che il vostro obiettivo è quello di creare il caos più assoluto. di fronte ad un'abrogazione sistematica di qualsiasi controllo, su chi entra o chi esce dal nostro Paese. Tutto questo è basato sulla retorica della confusione tra il soccorso e l'asilo. Lo dico ai colleghi, che sono un po' distratti: un conto è l'obbligo di soccorrere chi si trova in mare e rischia la vita e siamo assolutamente tutti d'accordo.

in automobile, trovo una persona che ha avuto un incidente, la raccolgo, la porto in ospedale, me ne prendo cura e poi quella persona viene a vivere nel mio letto. Non funziona così; non c'è un automatismo. Se una persona è stata soccorsa, ha diritto al soccorso non automaticamente all'asilo e a restare nel nostro Paese per tutta la vita; *(Applausi)* anche perché, Presidente - non le sfugge sicuramente - quelle persone non si trovano in mare per un caso, ma esiste un sistema ormai rodato, ben funzionante e molto efficiente per portare gente in Europa passando dall'Italia. Un sistema

altrimenti si perde di vista il quadro generale. Tuttavia, non si è ancora capito qual è il vostro piano, qual è il vostro progetto, a quale modello vi ispirate. Colleghi, sento parlare di modello tedesco,

il respingimento, l'espulsione o l'estradizione verso uno Stato, qualora esistano fondati motivi di ritenere - e qua c'è dentro tutto e niente - che ci siano rischi

mostruose nel ragionamento. È vietata l'espulsione di chiunque veda violato il rispetto della propria vita privata. Mi spiegate cosa vuol dire? persona, a casa sua, nel suo Paese, ha una legge che gli vieta di tenere il cane nel giardino, si considera mancato rispetto della vita privata e quindi ha il diritto di rimanere in Italia? Ancora, c'è il divieto di espellere chiunque non sia in perfetta salute psicofisica. Ciò vuol dire che se un soggetto trova uno psicologo che gli diagnostica una semplice depressione, automaticamente ha diritto di asilo perpetuo in Italia. O ancora, chi abbia processi in corso nel nostro Paese: praticamente chiunque gode del diritto di restare in Italia. Con il presente decreto-legge fate anche di più; immediatamente passate all'attivazione di tutto questo, ragion per cui il richiedente asilo ha diritto alla carta d'identità, a tutti i provvedimenti del *welfare* italiano, a tutto quanto spetta ai cittadini. Tutto ciò che una volta era riservato a determinate situazioni delicate e particolari, tutto ciò che una volta era collegato all'asilo per motivi seri oggi è sostanzialmente libero: chiunque viene, può restare. Peccato, però, che l'Italia è come una grande famiglia, come una grande casa; io in casa mia posso ospitare cinque, dieci persone; se stanno un po' strette, posso ospitarne anche 15 per un po' di tempo, se dormono a strati, col sacco a pelo sotto al tavolo; ma non posso ospitare tutti per sempre. Questo è il punto: non possiamo ospitare tutti per sempre. Abbiamo un dovere - e nessuno sta dicendo che questo dovere non debba essere rispettato - che è quello di soccorrere, ma torno a dire: avete preso coscienza di come funziona la rotta

vengono reclutate nei villaggi e viene loro raccontato che c'è un futuro fulgido in Italia; normalmente si tratta dei ragazzi più ricchi del loro villaggio, delle ragazze più belle venite in Italia, che è meraviglioso, intanto date 2.000 o 3.000 euro a chi vi organizza il viaggio. Questi ragazzi vengono strappati dai loro villaggi, vengono portati nei centri della Libia, normalmente vengono violentati e trattati da cani; dopodiché, dopo che sono rimasti lì per mesi, finalmente li portano a imbarcarsi su delle bagnarole malsicure e molti di quelli pagano con la vita affondando nel Mediterraneo

Questo è il futuro che avete in mente per il nostro Paese? Questo è il modello di accoglienza che avete in mente? Ebbene, noi a questo modello non ci stiamo! Noi a questo modello non ci assoggetteremo, per rispetto di quelle popolazioni. L'altro giorno parlavo con un caro amico vescovo

con chissà quali miraggi, con chissà quali promesse li state consegnando alla malavita, state mettendo le loro vite a rischio e tutto questo per che cosa? Qual è il modello che avete in mente? Ditecelo, cosa volete integrare. Volete l'integrazione? Siamo d'accordo. Ci sediamo a un tavolo e diciamo quante persone riusciamo a integrare. Le quote sono poche? Sono 30.000. Sono poche? Forse c'è posto per 35.000? Forse c'è posto per 40.000? Possiamo ragionare. Se pensate che ci sia spazio e se dimostrate che ci sia la modalità per integrare più di 40.000 persone all'anno, dimostratelo coi fatti, ma non potete permettere l'immigrazione clandestina in questo modo, perché questo significa uccidere i giovani, uccidere l'Africa che dite di voler tutelare *(Applausi)*, uccidere la speranza dei ragazzi di quei villaggi,

con attenzione la discussione generale e mi aspetto che dalla maggioranza venga una proposta. Non basta, infatti, portarli in Italia con queste modalità barbare; bisogna offrire loro una proposta seria. Mi riservo, in sede di replica,

Sospendo la seduta.

La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante

quattro ore e quaranta minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. La discussione avrà luogo nel prosieguo della seduta odierna per un'ora e quaranta minuti,

Alle ore 13,30 avranno luogo le dichiarazioni di voto con diretta televisiva e a seguire la chiama. *(Applausi)*.

Sono arrivato di corsa sulla sua sinistra e, all'altezza della sinistra dei banchi di Governo, ho ricevuto una fortissima gomitata all'altezza del cuore.

Dio ha voluto che alla violenza non reagissi con violenza. Mi sono spostato sulla parte destra dei banchi di Governo e mi sono diretto, come altri miei colleghi, verso i banchi di Governo.

non si debba ricevere violenza. E questo è il mio auspicio. Di solito non reagisco se una persona non è capace di intendere e volere. Nella mia carriera di sindaco mi è capitato di non reagire

in questa Aula più volte si è fatto riferimento ai principi fondamentali che presiedono ai decreti-legge. Da più parti si è sottolineata l'assenza dei requisiti di necessità e di urgenza. Consentitemi di fare qualche ulteriore, brevissima considerazione. La Corte costituzionale più volte ha precisato che i presupposti di necessità e urgenza devono anche essere assistiti dai requisiti di ragionevolezza e di non arbitrarietà.

il decreto è necessario per consentire il rispetto dei principi costituzionali e internazionali in materia. Ma se noi leggiamo il secondo dei decreti Salvini, scopriamo che già nei primissimi articoli vi è precisato che il decreto si applica salvo il rispetto degli obblighi internazionali. In realtà, in quest'Aula ho ascoltato più e più volte affermazioni che fanno parte di una narrazione falsa, costruita da una certa parte politica (da parte della sinistra, in particolare) a danno della Lega, una narrazione secondo cui addirittura i due decreti che si manifestano sullo sfondo trasformano in reato il soccorso dei migranti. Voi tutti sapete molto bene che questa affermazione è falsa, perché non si è davvero mai negato il soccorso a coloro che hanno bisogno. *(Applausi)*. Non una persona è stata lasciata in mare.

come dovrebbe essere normale in politica - ma un nemico, che voi screditate con una narrazione falsa. Questo decreto-legge serve a chiudere il cerchio per il vostro elettorato nei confronti di questa narrazione falsa. Voi in realtà state perseguendo un obiettivo politico legato alla soddisfazione del vostro elettorato a danno degli interessi del Paese: eliminando le sanzioni amministrative, voi rendete meno efficiente la gestione dei flussi migratori. Non ci dobbiamo dimenticare che la questione, ridotta all'osso, riguarda la gestione dei migranti economici. Nessuno ha mai inteso impedire la salvezza di coloro che scappano dalla guerra, di coloro che scappano dalla tortura o dalla persecuzione. il problema riguarda soltanto i migranti economici e vi devo ricordare che riguarda quei migranti che tentano di entrare illegalmente nel nostro Paese. Qui non è in questione l'accoglienza in quanto tale: è in questione la difesa della legalità. Quello che mi sembra incredibile è che non riesca a passare il principio che l'accoglienza, il soccorso e l'aiuto sono azioni che devono comunque iscriversi nel rispetto della legalità, della legge. I precedenti decreti servivano proprio a questo. Ora noi siamo anche più deboli nei confronti dell'Europa. È comprensibile che il Partito Democratico tenti quest'operazione. Mi sorprende assai di più la posizione degli amici del MoVimento 5 Stelle, che giusto due anni fa in quest'Aula difendevano questi decreti, anzi dicevano che erano necessari per rimediare al fallimento della precedente gestione. *(Applausi)*. Evidentemente adesso ritengono che si debba ritornare al fallimento. La verità amara è che c'è chi nella vita, per rimanere fedele a sé stesso, lascia un partito e c'è chi, per rimanere fedele a un partito, lascia sé stesso.

Grazie a tutti esame nasce da una osservazione del Capo dello Stato e da un appunto della Corte costituzionale su questi due punti si fonda. Poi, esso cerca anche di aggiungere qualche norma per garantire ancora meglio la sicurezza degli italiani e il rispetto dei profughi che nella nostra terra arrivano. La storia dell'evoluzione umana tutta è una storia di migrazioni. Non si ferma questo fenomeno con uno *slogan* o con delle norme che, alla luce dei fatti, si sono rilevate poco funzionali e neanche sicure per tutti. tutti. La posizione e la conformazione geografica hanno fatto nei secoli - e fanno - della nostra penisola, con le sue isole, anche le più piccole, un ponte nel Mediterraneo di congiungimento fra tre continenti: l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente asiatico; terra dove si sono incontrati e talvolta scontrati anche popoli, culture e culti; un grande zibaldone, oserei dire, e una straordinaria mescolanza millenaria, che ha dato impulso, nei secoli, a costumi, lingue e tradizioni ancora oggi diverse. C'è una cultura, ci sono dei costumi che ci uniscono e che esprimiamo nei più vari modi, finanche i tanti che simulano una gratuita e affettata idiosincrasia;

quando, invece di gioire o approfittare di un'occasione per mantenere il silenzio, qualcuno ha creato una *bagarre*

Detto ciò, tornando all'argomento in esame, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quella norma contenuta all'articolo 13 del decreto-legge n. 113 del 2018, che, di fatto, non riconosceva ai richiedenti protezione internazionale che ottenevano il permesso di soggiorno il diritto, ma anche il dovere -oserei dire - all'iscrizione anagrafica. Da tutti i punti di vista considerati, la norma censurata contraddice le finalità del decreto-legge n.113 del 2018, poiché la stessa non agevola il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto sicurezza stesso. La sicurezza la si ottiene con le regole chiare, con la possibilità di eseguire seri controlli per perseguire coloro che non rispettano le norme, anche le più elementari, e con la certezza della pena e la tempestività della stessa, come diceva un grande illuminista italiano. Elemento importante: il contesto attuale è anche cambiato rispetto a due anni fa. Quindi, con il decreto-legge in esame forniamo alle nostre Forze dell'ordine strumenti assai più efficaci di controllo per il rimpatrio degli irregolari. Abbiamo sempre creduto che la risposta più efficace fosse un sistema di accoglienza controllato, diffuso, efficiente e gestito in modo trasparente; punti tutti che, col presente decreto, vengono rafforzati. Ripetiamo, ancora una volta, che il tema è principalmente europeo e non dei soli Paesi di frontiera. Più in dettaglio, abbiamo dei percorsi per consentire un più facile monitoraggio ed evitare che quelle persone possano vagare per il nostro Paese e finire anche a delinquere. Evitiamo l'emarginazione, foriera di potenziali reazioni anche violente. Interveniamo sulle procedure di esame delle domande di asilo, con particolare attenzione verso le categorie particolarmente vulnerabili, come i minori, le donne in stato di gravidanza e gli anziani; ampliamo le competenze delle commissioni territoriali. Accorciamo i tempi di trattenimento per il rimpatrio degli irregolari, riducendo da centottanta a novanta giorni la permanenza nel nostro Paese e, soprattutto, ci rimettiamo in linea con le fondamentali norme di diritto internazionale. Noi non siamo per l'accoglienza indiscriminata, ma nemmeno per gli *slogan* su una materia così delicata e complessa:

il Governo ha lavorato proprio come Paese di frontiera con il nostro Ministro degli affari esteri una linea comune con la Spagna, la Grecia, Cipro e Malta. Circa 1.200 persone nel 2020 sono state rimpatriate dopo l'accordo con le autorità tunisine, che hanno dato la disponibilità a prevedere molti voli in più rispetto a quelli previsti. Consapevoli che la tratta di esseri umani non si sconfigge da soli e non la si può fermare in mare, né dentro i nostri porti, abbiamo rivolto al Governo tunisino una proposta di collaborazione che ha già avuto concreta attuazione. Non mi dilungo oltre. Ci sono anche norme più restrittive per i Daspo e per il contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti. In sintesi, sono tutte misure di buon senso, razionali, puntuali e soprattutto dettate da esigenze concrete, senza finalità demagogiche, sostenute da chi si oppone -come ho avuto modo di ascoltare che, senza entrare nel merito delle misure, si rifà a metodi faziosi e di semplice propaganda. Signor Presidente, Governo, colleghi senatori, l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita e disomogenea: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale; introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza; ridefinisce il ruolo del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale; pone un tema non chiaro di successione delle leggi nel tempo con ipotesi di retroattività riporta criticità diffuse. L'articolo 2 amplia l'ipotesi in cui l'impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla commissione territoriale non ha effetto sospensivo, allargandolo all'ipotesi di rigetto di domande presentate da persone sottoposte a procedimento penale penale o condannate per reati che costituiscono causa di diniego dello *status* di rifugiato. Si tratta di norma di coordinamento assolutamente necessaria in quanto, in caso contrario, la proposizione dell'impugnazione avrebbe prodotto l'effetto di congelamento dell'ordine di espulsione conseguente al rigetto proprio nei casi più gravi e di immediato accertamento. La possibilità di accertare immediatamente la sussistenza di tali condizioni dovrebbe condurre, anche in tal caso, nell'ipotesi più che probabile di richiesta di inibitoria degli effetti del provvedimento impugnato, una decisione monocratica di accoglimento o di rigetto, con modifica dell'attuale previsione dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, che contempla ben due pronunce collegiali, sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta di sospensione, con un *unicum* processuale, che non trova alcuna rispondenza con gli istituti in tema di inibitoria previsti dal codice di rito. Sembra indifferibile procedere verso l'individuazione di elementi diretti alla velocizzazione della fase del rito giurisdizionale dell'impugnazione dei provvedimenti delle commissioni territoriali. Ai sensi dell'articolo 35-*bis,* è bene ribadire che la richiesta di strumenti che consentono di rendere più agile e celere il rito è dovuta non soltanto - e ciò sarebbe bastevole -all'esigenza di affrancare i tribunali distrettuali da un numero insostenibile di procedimenti in materia di protezione, che costringono a sacrificare oltre ogni misura la tutela dei diritti dei cittadini, ma anche alla necessità di assicurare, in tempi ragionevoli e tali da essere conformi ai principi dell'articolo 111 della Costituzione, i diritti dei richiedenti asilo, nella consapevolezza che solo una tutela che intervenga in tempi celeri possa dirsi tale e sia in grado di proteggere l'effettività dei diritti fatti valere. Non sono stati valutati gli effetti applicativi della disciplina in esame con la finalità di approntare tutti gli strumenti legislativi utili che consentano di rendere più agile e celere il rito, anche mediante il passaggio dal rito collegiale al rito monocratico, al fine di poter impiegare nella decisione dei procedimenti tanti giudici quanti attualmente compongono il collegio, e di poter inserire in tabella anche i giudici onorari. Il provvedimento modifica norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, prevedendo la possibilità di automatica conversione del permesso di soggiorno per assistenza a minori in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il permesso di soggiorno per assistenza a minori, previsto dall'articolo 31, dispone che il tribunale per i minorenni possa autorizzare l'ingresso e la permanenza di un familiare del minore che si trova nel territorio italiano a precise e specifiche condizioni, ossia quando ricorrono gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore. La norma, oltre a prevedere tali condizioni in virtù dell'eccezionalità di tale permesso, che può essere concesso anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico, statuisce dunque che lo stesso debba essere rilasciato solo per un periodo di tempo determinato e comunque debba essere revocato quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio. È di tutta evidenza che tale permesso si configuri più come un'autorizzazione all'ingresso in Italia di natura eccezionale e contingente, proprio perché effettuato in deroga alle disposizioni previste dal nostro ordinamento che regolano l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale. La previsione della sua convertibilità in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro contrasta con la *ratio* dell'articolo 31, prestandosi a un uso strumentale della stessa. La mancanza di alcuna specifica condizione in merito alla effettiva capacità reddituale e al possesso di una idonea sistemazione alloggiativa, dove peraltro dovrebbe vivere il minore, e di una copertura sanitaria assicurativa espone ancor di più il nostro Paese a un incremento dei flussi migratori, attratti dalla prospettiva di poter facilmente ottenere un permesso di soggiorno in Italia. Già il Consiglio di Stato, con parere del 15 luglio 2015, si era espresso negativamente sulla convertibilità in permesso di lavoro di fattispecie di permesso di soggiorno da considerarsi un'eccezione, come nel caso di quello per assistenza a minori, rispetto all'impianto generale che poggia espressamente sulla programmazione dei flussi e sul sistema delle quote di ingresso. Non sono stati considerati - e concludo - gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative... ...di soggiorno per assistenza a minori di cui all'articolo 31, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il possesso in capo al richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.

il mio voto contrario all'odierno decreto-legge, per essere estremamente sintetica, si riassume in due ordini di motivi, uno prettamente politico e l'altro tecnico. Per addivenire alla cancellazione del decreto "Conte uno" ci si nasconde dietro i rilievi avanzati dal Presidente della Repubblica, non per migliorare l'impianto originario del cosiddetto decreto Salvini, ma solo per mostrare uno scalpo da esibire quale prova di fedeltà ai propri alleati. *(Applausi)*. non ricordare che votammo quel decreto-legge convintamente. Anzi, qualcuno in maniera colorita motivò il sì sostenendo che sarebbe servito a ridurre le corse dei taxi del mare. Ma non solo: si disse che il sistema dell'accoglienza diffusa era un'esperienza fallimentare. Bene, io continuo a credere che il sistema riproposto era e sarà costosissimo e inefficace. Appare poi ancora più disarmante la resa alle ONG, che in sostanza godranno di una patente di immunità. Nel nuovo testo unico sull'immigrazione e sui flussi di ingresso di stranieri in Unione europea si dispone che, in caso di mancata pubblicazione della programmazione triennale, il Presidente del Consiglio possa prevedere con proprio decreto. Sembrerebbe che, indipendentemente dalla necessità di manodopera straniera, l'Italia sia vincolata ad accogliere immigrati. immigrati. Vorrei comprendere verso chi abbiamo questo obbligo. Per concludere, Presidente, si prevede massima discrezionalità al Presidente del Consiglio nell'accogliere, ma nello stesso tempo l'abolizione della discrezionalità dei questori nella valutazione per la revoca o il rifiuto del permesso di soggiorno. Forse, chiedere ad un questore perché a volte si

aiuterebbe a capire perché non bisogna votare questo nuovo decreto-legge.

il provvedimento in discussione è sbagliato nel merito ed è sbagliato nel procedimento. È stato detto prima chiaramente che nel merito è sbagliato perché riapre in maniera indiscriminata i porti e ridà benzina alla mangiatoia e agli affari che ci sono intorno all'immigrazione clandestina. *(Applausi)*. È sbagliato nel procedimento, perché non sussistono i presupposti di necessità e di urgenza per la decretazione d'urgenza. Ricordiamo, è sbagliato anche nel contesto, perché questo provvedimento cade nel pieno di una pandemia mondiale che i nostri figli leggeranno sui libri di storia,

le partite IVA, gli imprenditori sono in ginocchio, questo Governo pensa a rivedere i decreti Salvini *(Applausi)*. nell'interesse dell'Italia, ma perché è guidato da due bestie che in politica non devono guidare una scelta di governo: il furore ideologico e l'accanimento personale. Questo è alla base di questo decreto-legge. voglio rivolgere una domanda, con rispetto ma anche fermezza, ai colleghi del MoVimento 5 Stelle: cari colleghi, sapete cosa vi accingete a votare? Sapete che quello che vi accingete a votare è l'esatto contrario di ciò che avete votato circa due anni fa? Sapete che state facendo l'esatto contrario? Avete detto poco tempo fa che la cura migliore per gestire l'immigrazione era regolamentare gli accessi, chiudere i porti, regolare in maniera intelligente gli accessi sul nostro territorio. Oggi siete per l'immigrazione clandestina e per l'immigrazione allegra. *(Applausi)*. Fate il contrario di quello che avete fatto prima, ma vi è di più ed è successo a Catania pochi giorni fa: rinnegate anche ciò che avete eseguito; quell'ex ministro, un vostro collega, di cui noi ricordiamo benissimo il nome perché abbiamo ottima memoria, Toninelli, ha rinnegato ciò che con vanto diceva di aver fatto nell'interesse dell'Italia. Ecco qui una differenza: a Catania, grazie a Dio, a differenza del vostro collega, si è visto un uomo che, con vanto e orgoglio, ha ribadito ciò che ha fatto nell'interesse dell'Italia e coordinandosi con una volontà collegiale di quel Governo. Per concludere, signor Presidente, la differenza tra noi e voi si può riassumere in un contegno: per noi il Viminale è

Pochi giorni fa la procura della Repubblica di Potenza ha eseguito delle ordinanze di custodia cautelare per combattere tutto il *business* che ruota intorno all'immigrazione clandestina.

due presunti delinquenti - l'imprenditore agricolo che utilizzava questi contratti fasulli e l'intermediario - l'imprenditore agricolo diceva che pensava che i controlli dell'Ispettorato del lavoro fossero dovuti a qualche spia. L'intermediario diceva: no, purtroppo non è qualche spia, questa è la mano del ministro Salvini, che mira a combattere l'immigrazione clandestina. Questo significa, leggendo le carte della Procura della Repubblica dalla stampa, che quello era uno strumento per far entrare sul nostro territorio soggetti pericolosi per la nostra Nazione.

rischiate di far perdere tempo all'Italia, ma non pensate di fermarci, perché non ci riuscirete. Signor Presidente, con la conversione del decreto-legge in tema di immigrazione e sicurezza si interviene sulla normativa nazionale perché, tra le altre cose, si allinei al rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale. L'intervento fondamentale del provvedimento è la previsione che il rifiuto e la revoca del permesso di soggiorno non possano essere adottati quando ricorrano seri motivi derivanti dal rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. Questo, come altri passaggi, risponde anche a quanto espresso dal presidente della Repubblica Mattarella in sede di emanazione del decreto sicurezza nell'ottobre 2018. Nella fattispecie, il Presidente richiamava la necessità che in materia restassero fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. Colleghi, nessuno può morire o essere torturato a causa del proprio orientamento sessuale, della religione che professa o del colore della pelle, ma soprattutto - lasciatemelo dire - nessuno merita di morire perché qualche partito ci possa costruire sopra una campagna elettorale. Usare l'odio e la paura per raccogliere *like* e racimolare consensi è quanto di più basso la politica possa concepire. A proposito di odio, vorrei manifestare la nostra solidarietà al collega Danilo Toninelli, che è stato sottoposto a un'aggressione mediatica basata su indegne e pilotate *fake un'aggressione mediatica basata su indegne e pilotate *fake news*. *(Applausi. Commenti)*. Le conseguenti minacce che ha ricevuto via *social* sono un preoccupante segnale di un crescente clima di odio. Presidente, mi permetta una precisazione. A chi accusa il MoVimento 5 Stelle di aver cambiato idea sulle politiche migratorie rispondo con sincerità. Oggi siamo sollevati di poter modificare questi decreti-legge, perché non ci hanno mai pienamente convinto. *(Commenti)*. Li votammo solo nel rispetto di un accordo di Governo, ma come temevamo e segnalammo - le evidenze lo hanno dimostrato le disposizioni dei decreti sicurezza sono inefficaci. Nel lungo periodo quei provvedimenti si sono rivelati per quel che erano: degli *spot* propagandistici inutili. A proposito della differenza tra chi fa *spot* e chi invece fa i fatti, vorrei ringraziare il presidente Conte, il ministro Di Maio e l'intero Governo per il lavoro che ha portato alla liberazione dei 18 pescatori italiani. Sì, ci piacciono i fatti, come anche il progetto di formazione agricola per i giovani del Ghana inaugurato un anno fa dal Presidente del La posizione del MoVimento 5 Stelle in tema di immigrazione è diversa dalla vostra. Noi siamo per un approccio pragmatico e non ideologico, che giudica le soluzioni non perché sembrano di sinistra o di destra, ma perché funzionano o non funzionano alla prova dei fatti i fatti hanno dimostrato che il traffico illegale di migranti non si è fermato con le modalità proposte dalla destra. Possiamo dirlo una volta per tutte: la Lega ha fallito *(Commenti)*, ha fallito nell'unica battaglia che contraddistingue la sua politica una politica di antagonismo che vuole alimentare una guerra tra poveri, voluta e studiata per creare conflittualità tra i migranti e quegli italiani, in difficoltà economica, vittime delle politiche di *austerity* che nessun Governo, prima di quello attuale, era riuscito a far cambiare a Bruxelles. Il nostro obiettivo deve essere quello di coniugare un'immigrazione sostenibile con la pacificazione sociale e non di seminare paure, nascondendosi dietro la bandiera di quell'Italia che un tempo loro stessi volevano dividere. Salvini, al di là dei suoi *slogan* da difensore delle patrie frontiere, ha fatto i suoi *show*, fermando qualche nave da soccorso delle ONG carica di pericolosissimi naufraghi, dimenticandosi dei cosiddetti sbarchi fantasma,

A chi continua a ripetere che nell'ultimo anno gli sbarchi sono triplicati, ricordiamo che per cortesia. FERRARA *(M5S)*. A chi continua a ripetere che nell'ultimo anno gli sbarchi sono triplicati, ricordiamo che fino a due mesi fa i decreti Salvini erano ancora in vigore, a dimostrazione che il fenomeno non si ferma con un decreto. L'ex ministro dell'interno aveva promesso di rimpatriare tutti gli immigrati irregolari presenti in Italia. Vi sembra che sia successo?

Presidente, colleghi, la realtà è che Matteo Salvini ha fatto solo il bullo sulla pelle della povera gente Brandendo il rosario ha portato avanti una dialettica di odio, opposta a quell'immagine di carità cristiana e di compassione che il rosario dovrebbe simboleggiare. Almeno in questo tempo di Natale si dovrebbe rileggere la parabola del buon samaritano. Lui si è illuso di poter costringere l'Europa a fare la sua parte, ma ha ottenuto l'effetto contrario. Oggi l'Italia, invece, non solo partecipa attivamente, ma, grazie al grandissimo lavoro del presidente Conte, sta cambiando l'Europa anche su questo, preparando il terreno per il superamento degli anacronistici regolamenti di Dublino votati dalla destra. Questo è ciò che il MoVimento 5 Stelle chiede da sempre in tema di immigrazione, insieme all'istituzione di canali legali e sicuri di ingresso in Europa per i richiedenti asilo. È dalla scorsa legislatura che sottolineiamo quanto sia importante affrontare le cause profonde delle migrazioni questo significa puntare sulla cooperazione internazionale, per contrastare povertà e disoccupazione, allo scopo di garantire ai giovani di quei Paesi il sacrosanto diritto di costruirsi una vita e una famiglia vicino ai loro affetti, senza essere costretti ad andare a cercare fortuna altrove. Presidente, dobbiamo evitare l'ipocrisia di chi con una mano dà e con l'altra toglie. È inutile fare attività di cooperazione, se si continuano a tollerare forme di neocolonialismo e di sfruttamento predatorio delle risorse naturali, finanziarie e e umane del Continente africano. Concludo dicendo che oggi, con il provvedimento in esame, vogliamo conciliare in modo più equilibrato accoglienza e sicurezza, rispetto del diritto internazionale e i principi fondamentali della Costituzione italiana e vogliamo dimostrare che, più dei consensi elettorali, ci interessa tutelare la sacralità della vita umana e una giusta coesistenza.

n. 87, contenente norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, ho l'onore di comunicarLe che il Collegio di questa Corte Suprema di Cassazione, appositamente convocato, ha eletto in data odierna la dottoressa Maria Rosaria

Grazie a tutti

ma visto che tanto ve ne fregate bellamente di ciò che state facendo, cerco di argomentare in altro modo. Pertanto utilizzerò il tempo che, fortunatamente, la democrazia ancora mi concede, per dirvi ciò che penso del vostro decretino, lontano anni luce dal contesto che gli italiani stanno vivendo. Sabato mattina ero a casa e, mentre la TV passava in diretta le notizie da Catania, tra un ricordo strano e un «non so» di Toninelli, mi chiedevo come un ex Ministro possa arrivare a tanto. Pensavo a quella leggerezza e pensavo al decreto sicurezza, che oggi siamo qui a discutere. quando abbiamo scritto i decreti Salvini, lo abbiamo fatto con tutti voi. *(Applausi)*. Li avete addirittura emendati e il vostro attuale Capogruppo era il mio Presidente di Commissione: insieme a lui li abbiamo emendati e li abbiamo rivotati successivamente in Vi siete espressi favorevolmente per ben tre volte e oggi cambiate il decreto-legge come se nulla fosse, con tutta questa semplicità. Non sono un medico - ci mancherebbe altro - ma credo che, in medicina, questo sia un grave disturbo del comportamento *(Applausi)* e abbia un nome ben preciso. Non voglio pensare che questa sia solo ignoranza, ma voglio darvi un alibi. Nella stesura dei decreti-legge sapevate benissimo di mettere, con noi, nero su bianco, la parola fine all'invasione clandestina e ci eravamo anche riusciti. Oggi, dopo mesi, grande capriola: chissà cosa è successo? Un giorno ce lo spiegherete o forse l'abbiamo già capito e lo sapete benissimo anche voi. Forse era meglio se foste andati avanti ad occuparvi di TAV. No, scusate, ho sbagliato esempio. Forse era meglio il MES? Anche quello però è andato male.

no, accidenti! - ma qualcosa deve sempre andare storto, eh! Qualcosa va sempre storto, chissà perché. La verità è questa, carissimo amico mio; la verità è che siete entrati verginelle qui dentro e state uscendo pornostar! *(Applausi).* Questa è la verità! Forse è meglio che torniate a "cazzeggiare" sul *web*, almeno lì non fate danni, amici miei! Almeno lì non fate danni!

Magari, poi, ci sarà Di Maio che inventerà l'indagato zero, così risolviamo anche quel problema, Presidente. *(Applausi).* Ma torniamo a noi. Vi voglio citare i numeri, perché sono stati i numeri a parlare, non le chiacchiere dette così, tanto per parlare. quindi, appena entrato in vigore il decreto-legge Salvini, durante l'immediata attuazione dello stesso siamo passati - pronti, via! - da 1.654 a 757 sbarchi; i cadaveri recuperati in mare passano da

e mai una risposta mi è stata data: chi sono veramente gli assassini, Presidente *(Applausi),* quelli che salvano le vite e si battono per la sicurezza e la difesa dei confini interni ed esterni oppure quelli che lasciano morire donne e bambini in mezzo al mare, alimentando il *business* dell'immigrazione clandestina? Vedete, voi avete solo una grande voglia di smantellare i decreti-legge Salvini per ricominciare la tratta di esseri umani nel Mediterraneo. Mi rivolgo agli amici del PD: ma quanti amici degli amici ancora dovete fare ingrassare sulle spalle degli italiani prima di fermarvi? *(Applausi)* Continuiamo, continuiamo. Magari, importate malati di Covid che nessuno controlla, nessuno blocca, nessuno cura, e poi, come nulla fosse, li ricollochiamo magari nei paesini, obbligando i sindaci ad accoglierli, come se quello fosse il problema primario. Il problema primario oggi sono i nostri nonni che affrontano la morte in solitudine e nel silenzio delle istituzioni; li stiamo lasciando soli: questi sono i problemi della gente. *(Applausi)*. Poi, sarà colpa dei Presidenti delle Regioni, sarà colpa della sanità regionale, dei sindaci, ma mai del Governo: l'Esecutivo in tutto ciò non avrà mai una colpa perché la responsabilità è sempre un peso grosso da portarsi dietro. Concludo, Presidente, perché penso di aver esaurito il tempo Siate coerenti almeno con voi stessi, amici 5 Stelle; rispettate ciò che avete fatto la prima volta, perché quella era la strada giusta. Non cadete in questa triste tentazione che vi stanno mettendo di fronte; state sbagliando completamente. Ciò che dovevate fare era seguire noi in questa partita e non salvare le poltrone e seguire una battaglia che non è vostra; è una battaglia del Partito Democratico, non vi appartiene. State schiacciando con un piede la gola di una tigre. State molto attenti, perché un giorno arriverà il momento di togliere quel piede, ma non sarete voi a deciderlo.

Signor Presidente, questo è un momento molto importante. Come è stato detto, sicuramente

in esame rimette finalmente le cose a posto dopo i tanti danni fatti sulla pelle delle persone, dopo i tanti fantasmi lasciati sul territorio italiano senza un'identità Grazie a tutti dando manodopera al lavoro nero e all'illegalità. Questo chiaramente è accaduto per la mancanza di iscrizione alle anagrafi. Ci siamo rimessi sui giusti binari della correttezza costituzionale, del rispetto degli obblighi internazionali e delle convenzioni dei diritti umanitari e delle leggi, perché non basta enunciare i principi nei capoversi se poi si contraddicono pesantemente nelle disposizioni e nei fatti. Vorrei però elencare punto per punto quello che troviamo nel decreto-legge, perché si è fatta molta mistificazione, quindi è importante dire cosa è stato fatto.

che tante buone pratiche ha messo in atto e dove vengono inclusi anche i richiedenti asilo, che erano invece esclusi dai cosiddetti Abbiamo il ritorno all'iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, che è l'unico modo per sapere chi è sul nostro territorio e per non lasciarlo nelle mani della criminalità. Si ampliano le casistiche del divieto di allontanamento, per cui non si può disporre l'espulsione e il respingimento di uno straniero oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni politiche e sociali e neanche per l'orientamento sessuale e l'identità di genere (grazie a un emendamento approvato o per seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Questa precisazione, per un inciso che era stato abrogato dal decreto-legge n. è stata voluta alla Camera; si tratta di un richiamo importante esplicito al rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano. Si deve poi tener conto che un allontanamento dal nostro territorio nazionale non deve comportare una violazione del diritto e del rispetto della vita privata e familiare dello straniero. Sono inoltre

il ridimensionamento delle multe sproporzionate per le organizzazioni non governative e l'applicabilità delle multe solo dopo procedimento giudiziario, che non trova però applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso. chiaramente, nel rispetto delle regole, come è ovvio. Ancora, nell'ottica che per sconfiggere il traffico di esseri umani e l'immigrazione illegale occorre creare canali di accesso legali, vengono superati i limiti temporali e numerici del cosiddetto decreto flussi (l'ultimo è del 2016), che dovrebbe ogni anno regolare i flussi d'ingresso di stranieri per motivi di lavoro. Solo così si ha immigrazione irregolare. E si delineano interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale, l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, prevedendo, nel contempo, ove possibile, qualunque strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. Si interviene Si interviene ancora sulla convertibilità di alcuni permessi di soggiorno in permesso di lavoro per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi, per assistenza minore e per cure mediche dovute a gravi condizioni psicofisiche e gravi patologie. Anche quest'ultima è una voce voluta dalla Camera, ossia dal Parlamento. Si interviene sulla competenza a limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, sopprimendo l'attribuzione che il cosiddetto decreto-legge Salvini poneva arbitrariamente in capo al Ministro dell'interno; e si sopprimono le disposizioni sanzionatorie per il comandante della nave che violi il divieto di ingresso nel mare territoriale nonché la relativa confisca e distruzione delle imbarcazioni. Si prevede, infine, l'allargamento dei motivi per permessi speciali di soggiorno. È stato fatto tutto? No, ora bisogna superare la cosiddetta legge Bossi-Fini. Serve una riforma della legge sulla cittadinanza e sull'immigrazione ed un'efficace modifica UE del Regolamento di Dublino. Quindi, c'è da lavorare.

del Governo, colleghi, la cosa più triste di questa giornata, che è cominciata con la bella notizia dei pescatori che tornavano in Italia, è l'insondabile sensazione che abbiamo tutti noi dell'inutilità di un lavoro consegnato già in premessa alla fiducia, e come tale immodificabile. Noi stiamo parlando intorno ad un oggetto che non sarà possibile modificare nemmeno di un attimo. La cosa ancora più triste è che la prossima settimana ci aspetterà la legge di bilancio e poi il cosiddetto decreto Calabria: e sarà la stessa cosa. E la settimana scorsa era ugualmente la stessa cosa. La tristezza nasce dal fatto che tutto il nostro dibattito non riuscirà a migliorare di una virgola un provvedimento che probabilmente contiene, come è normale, alcuni aspetti positivi, ne contiene altri sicuramente problematici e ne contiene alcuni che, per una parte di noi, non sono condivisibili. Ma il problema è l'inutilità del lavoro; è questo sistema che è invalso in questa seconda parte di legislatura, per cui siamo un sistema monocamerale a corrente alternata. Non è possibile. Questa è, nei fatti, una riforma di stampo costituzionale che infrange quello che nell'orizzonte dei Padri costituzionali è un sistema bicamerale. La nostra è una Repubblica parlamentare che ha un suo andamento strettamente legato all'aspetto bicamerale. Noi stiamo mortificando la prima parte attraverso l'insistenza sistematica, costante e continua di decreti e DPCM, stiamo mortificando la seconda parte attraverso questo sistema di Camere ad andamento alternato. Non so se ci si rende conto; non so se chi ci ascolta o la stampa domani sarà in grado di rivelare ai cittadini il *vulnus* che si sta creando: creando: il vero *vulnus*, oggi come oggi, è l'inutilità del lavoro che, in modo alternato, una Camera e l'altra fanno. La *bagarre* di oggi ci ha fatto vivere per tre o quattro ore in sospensione. Che cosa dirà la Capigruppo? Che cosa succederà? Che cosa poi noi potremmo fare? Come ci dovremmo regolare? Tutto ciò è una tale mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento la dice lunga. Come possiamo rispettare noi i migranti che arrivano se non siamo capaci di rispettare nemmeno il nostro lavoro? E qui entro nel vivo del decreto-legge.

tutto ciò lo sappiamo benissimo perché chi di noi è in Parlamento da più di una legislatura sa che il dibattito si ripete tutte le volte, ma poi non ci sono i modi - i famosi decreti attuativi per renderlo possibile e realizzarlo. Mi sembra meravigliosa la possibilità che possano venire a studiare in Italia. Tutti voi sapete che tutte le università si sono attrezzate con corsi in lingua inglese per attrarre studenti stranieri, per ottenere che l'internazionalizzazione possa diventare un elemento efficace di arricchimento,

Abbiamo detto che possiamo accogliere - lo diceva la collega che ha parlato prima - le persone affette da patologie gravi, ma già lo facciamo. Tutti sanno, per citare solo un ospedale, che il Bambino Gesù è aperto ad accogliere i bambini in situazioni drammatiche e - cosa da non dimenticare - sulla base del nostro sistema sanitario ciò avviene in condizioni di totale gratuità.

se non ci fosse questa logica di apertura, anche se dopo si incorre in incidenti di percorso? Abbiamo visto quanto è accaduto recentemente tra la Juve e l'Università per stranieri di Perugia.

non la prima generazione. Il nostro vero problema è riuscire a trasmettere alla seconda generazione quel livello così profondo di integrazione che li faccia sentire italiani. E per farli sentire tali c'è tutta una serie di condizioni che vanno messe. Penso alla casa, che non è il centro di accoglienza o questi famosi luoghi dove arrivano e da cui fuggono perché non rispondono alle condizioni attese di umanità e alle promesse. Hanno bisogno di lavoro, ma tutti noi stiamo vivendo nel terrore annunciato che non deriva tanto dalla terza ondata del coronavirus, ma dalla drammatica situazione della disoccupazione, dell'inoccupazione e dei licenziamenti. È inutile che ci venga detto tutte le sere che le situazioni miglioreranno. Sappiamo tutti che il PIL è in caduta libera. Ce l'ha ricordato pochi giorni fa anche il famoso Draghi, che, quando è stato a Rimini, ha parlato di debito buono e di debito cattivo, e ha letto il debito buono in termini di investimento e, quindi, di occupazione che si crea. Lui stesso però due giorni fa ha detto che l'occupazione non si potrà creare per la semplice ragione che nel manifatturiero abbiamo perso moltissimi colpi e per la mancanza delle grandi infrastrutture, che sono quelle che rendono possibile l'occupazione e che non ci sono. Sappiamo che i migranti che arrivano spesso si riducono a fare i lavori che gli italiani non vorrebbero fare, ma è semplicemente questione di un tempo minimo perché anche loro non vorranno fare quei lavori se non interverremo implementando la dignità e il riconoscimento economico e sociale di queste attività.

Oggi noi saremmo dovuti intervenire per dire come fare questo, come garantire certe tutele. Sapete che nella legge Zampa - lo dico se qualcuno dei colleghi nella precedente legislatura non l'avesse letta - si dice che ogni bambino che arriva in Italia non accompagnato ha diritto ad un tutore, che non significa ovviamente adozione o affido, ma è una presa in carico? Voi avete visto i minori non accompagnati e i tutori? Ci sono forse tutori per tutti questi bambini? Non ci sono, spariscono

la strada è quella dello spaccio. Alla Camera, in questo momento, tra le tante questioni che stanno studiando nella legge di bilancio, c'è anche la legalizzazione della droga.

Invece, poiché non serviva a nulla questo dibattito, perché tanto il decreto era già congelato, non ci siamo interrogati sul se fare, ma nemmeno sul come fare ed è una grande tristezza perché vuol dire che siamo sempre al punto di partenza. Signor Presidente, dopo una lunga opposizione alla Camera e nelle Commissioni del Senato, oggi il Parlamento prende atto che il Governo, utilizzando come pretesto indicazioni limitate giunte dalla Presidenza della Repubblica su alcune norme introdotte nei cosiddetti decreti sicurezza, ha deciso, senza alcuna ragione, di stravolgere la legislazione in tema di immigrazione e sicurezza, a conversione quello che passerà alla storia come il decreto clandestini, introducendo norme del tutto estranee rispetto alle cosiddette indicazioni, senza che vi sia alcuna esigenza rispetto alla pandemia mondiale e alla crisi sanitaria ed economica che sta vivendo il Paese. Sebbene sia difficile da credere, è assurdo che tutto ciò avvenga con il benestare del MoVimento 5 Stelle, la parte più numerosa della maggioranza, quella parte che solamente un anno fa con il proprio voto favorevole aveva convintamente adottato gli stessi provvedimenti che oggi si vogliono rinnegare e smantellare. Chissà se anche in questa occasione ci si vuole rifugiare in un «Non ricordiamo»? Saremo noi a ricordarvelo e saranno gli italiani a ricordarselo. L'unica emergenza di cui si dovrebbe discutere è la pandemia globale, che ha colpito il mondo intero e il nostro Paese e la crisi economica e sociale che ne è conseguita e non ha precedenti dagli anni del Dopoguerra. Dovremmo discutere di questo, di quali provvedimenti il Governo intende adottare per far fronte a quanto sta avvenendo nel mondo reale e a supporto dei cittadini italiani, ricordando che se siamo in quest'Aula è per rappresentare i loro interessi. Gli italiani vorrebbero sapere, dopo mesi di restrizioni e sacrifici, cosa potranno fare il giorno di Natale; se potranno incontrare nuovamente i loro cari o se, invece, ciò non sarà loro consentito. Per questa maggioranza, evidentemente, tutto questo non è prioritario. Appare incredibile, ma, evidentemente, l'urgenza di questa maggioranza è agevolare ingressi illegali nel nostro Paese, rivedendo quelle stesse norme che hanno, dopo anni di pessima gestione di flussi migratori, restituito al Paese delle regole capaci di garantire sicurezza interna di limitare le partenze dalle coste dei Paesi del Nord Africa e, di conseguenza, gli ingressi nel nostro Paese e le dolorose morti nel Mediterraneo.

da coronavirus, il Parlamento non sta discutendo dell'opportunità di riconoscere protezione internazionale a soggetti che fuggono da Paesi coinvolti in conflitti armati (fattispecie da tutti riconosciuta suscettibile di salvaguardia). Al contrario, si sta discutendo di come riaprire il Paese a flussi incontrollati e irregolari di immigrazione, che con l'attuale Governo, è bene ricordarlo, risultano già quadruplicati rispetto a quelli registrati quando era ministro Salvini. Si sta introducendo l'impossibilità di porre un limite all'ingresso, al transito e alla sosta di navi ONG che abbiano svolto operazioni di soccorso in mare, diminuendo drasticamente le sanzioni a seguito di inosservanza del divieto di transito in acque territoriali italiane. Di fatto, si sta portando a compimento quel processo di degenerazione della gestione di flussi migratori, cui stiamo assistendo dall'insediamento di questo Governo e del ministro Lamorgese Trovo deplorevole che, in questa fase drammatica, la priorità dell'Esecutivo sia di aumentare in maniera esponenziale il numero dei permessi di soggiorno per gli immigrati, ampliando le casistiche legittimanti

si vanno ad inserire una serie di norme sconsiderate, tra cui la riduzione dei termini per la concessione della cittadinanza e il divieto di espulsione dei soggetti che paventino discriminazioni legate all'orientamento sessuale, generando confusione sulla loro applicabilità e lasciando alla discrezionalità di magistrati una gestione farraginosa e poco chiara, cui prevedo seguiranno un'infinità di ricorsi.

Avevamo chiuso il capitolo dell'invasione clandestina due anni fa, quando avevamo approvato i decreti Salvini, ma, in realtà, sarebbe stato troppo intelligente e normale lasciare le cose come erano, perché funzionavano.

Siete pionieri del caos. Le vostre radici anarchiche, da centro sociale, ogni tanto riaffiorano. È un po' la vostra natura. Così, quando approvate una buona legge, voi vi sentite più o meno come un pinguino nel deserto: siete a disagio, sudate, non state per Se cancellerete i cosiddetti decreti Salvini farete entrare in Italia persone di cui non si sa assolutamente nulla e che, per la maggior parte, come sapete benissimo, fuggiranno poi dai centri di identificazione, riversandosi per le nostre strade.

Persone di cui non conosciamo la reale provenienza, per le quali non c'è stato alcun tipo di controllo sulla loro identità, sulla loro eventuale pericolosità sociale, sul loro effettivo *status* di rifugiati o - figuriamoci - sulle loro competenze lavorative. Bravissimi, la malavita ringrazia sentitamente per la fornitura di manodopera a bassissimo costo. *(Applausi)*. Ah, no, scusate, un prezzo ce l'ha ed è il prezzo dei sogni di quella gente su cui poi voi andrete a lucrare con le vostre ONG. ONG. È abbastanza ovvio infatti che il tessuto sociale ed economico che abbiamo in Italia in questo momento non può assorbire qualunque flusso migratorio. Solamente voi però non riuscite a capire questa cosa. Quanto sarebbe bello poter permettere agli italiani di votare per dire cosa pensano di come il Partito Democratico ha gestito l'immigrazione in Italia da Monti ad oggi.

l'opinione pubblica in un senso ipocrita e buonista, per giustificare il *business* dell'immigrazione. Era la mangiatoia dei benpensanti. Servirebbero punizioni rapide e severe per i trafficanti di esseri umani, ma voi, ancora una volta, con il vostro agire negate l'evidenza. I nostri decreti sicurezza prevedevano infatti misure atte a migliorare l'efficacia dell'azione delle Forze dell'ordine; erano norme operative ed utili per chi fino a ieri si trovava ingessato nella propria azione di controllo del territorio per la mancanza di queste leggi, ma anche e soprattutto per la mancanza di uno Stato schierato al loro sostegno senza se e senza ma. Siamo al paradosso. Smantellate una norma e, per giustificare questo scempio, cercate di usare scuse come i vuoti normativi. È chiaro a tutti che l'unico vuoto che esiste è quello della vostra azione politica. Dove eravate in tutti questi anni in cui il territorio implorava un aiuto, un intervento, una legge a favore dei cittadini onesti? E soprattutto dove siete oggi, cosa fate oggi nel momento in cui tutte le energie dovrebbero essere concentrate per aiutare le attività produttive, i bar, i ristoranti, gli hotel e le aziende, sacrificate per gestire l'emergenza Covid? Cosa state facendo? Approvate una legge che rende le nostre strade ancora più insicure di quanto siano in questo momento. Per noi, in Italia, non c'è spazio alcuno per clandestini e criminali; per noi i diritti degli onesti vengono prima di quelli dei delinquenti. Strano? Avete creato le condizioni ideali per far sbarcare persino assassini e terroristi; ricordatevelo perché è un'onta che non si lava facilmente. Dovreste scusarvi, dimettervi e nascondervi per la vergogna. Invece ricominciate a porre le basi per una nuova invasione di massa,

State creando un esercito per la malavita. Davvero la vostra poltrona vale più della vostra credibilità. Ne avete ancora qualcosina, un briciolo, un pizzico? *(Applausi)*. Presidente, in conclusione, a causa vostra ci saranno nuovi rischi per la sicurezza e la salute pubblica e altri altri soldi per l'accoglienza verranno chiesti agli italiani. Questa sarà l'ennesima scelta di bandiera odiosa, insostenibile e tanto lontana dalla realtà, quanto i *radical chic* che dai loro palazzi d'avorio promulgano l'ennesima porcata a danno dei cittadini italiani onesti. Prima o poi però

Governo, lasciatemi una premessa: siamo felici, felici, felici che i 18 pescatori di Mazara del Vallo siano stati liberati e per questo ci uniamo al coro dei ringraziamenti alla nostra *intelligence*, che ancora una volta è riuscita a risolvere un caso all'apparenza disperato. Quindi buon Natale a loro e buon Natale alle loro famiglie. Ma veniamo a noi. Mi sembra surreale, anzi, è surreale che oggi, 17 dicembre 2020, in un momento come questo in cui l'Italia intera sta vivendo con il fiato sospeso, grazie - si fa per dire - a un Governo che non è in grado di dare tranquillità, perché totalmente inadeguato e confuso: in un momento come questo, in cui l'Italia sta vivendo uno dei peggiori periodi della sua storia contemporanea, con in corso una crisi a tutto campo

in un momento in cui i cittadini non sanno cosa riserverà loro il futuro, a partire da quello prossimo, che vedrà a partire da quello prossimo, che vedrà le famiglie divise a Natale, famiglie come quelle del mio territorio bergamasco, che hanno perso già in maniera straziante i loro cari; in un momento in cui il Governo non è in grado di realizzare un progetto che vada al di là del giorno per giorno, in un *carpe diem* snervante; in un momento in cui pende sulla testa dei cittadini la spada di Damocle dell'apertura dei licenziamenti, della chiusura delle attività

collaborare insieme alla stesura di un piano progettuale di investimenti per poter usufruire del *recovery fund*, che è condizionato alla creazione di un progetto di visione per garantire la sopravvivenza sostenere la ripartenza del Paese durante e dopo la pandemia (e potrei andare avanti all'infinito), su cosa questo Governo fa lavorare il Parlamento? Lavorare Lavorare per modo di dire, perché ormai il Parlamento lavora sì giorno e notte, ma come un moderno Sisifo, chiamato solo a votare scandalose e snervanti fiducie, ad esempio su un provvedimento come il decreto immigrazione-*bis* PD, da convertire in legge secondo caratteri di eccezionalità e di urgenza che non sussistono.

lungi da noi il pensiero di lasciare indietro chi soffre, di non voler aiutare i più sfortunati; ma noi lo vogliamo fare *cum grano salis*, creando tutte le condizioni necessarie per gestire al meglio un fenomeno che potrebbe diventare inarrestabile se non lo si affronta in maniera seria e coinvolgente, partendo dagli accordi bilaterali a livello europeo, ma anche mondiale, passando dal mettere in atto ogni iniziativa mirata ad aiutare concretamente le persone a crescere e prosperare nel loro Paese (il famoso piano Marshall, che adesso forse serve più all'Italia che all'Africa), ma soprattutto a non essere turlupinate e prese in giro. Questa è la serietà, proprio per il profondo rispetto della dignità della persona umana e dei diritti fondamentali di ogni singola persona, secondo il medesimo concetto che stiamo cercando di far passare da noi in Italia, soprattutto oggi, in questo momento difficile: l'assistenzialismo fine a se stesso non serve a nulla, se non è affiancato da interventi e azioni concrete di investimento rispetto alla realizzazione di condizioni idonee a creare lavoro e rendere autonome le persone. Bisogna agire, di fronte all'aumento degli sbarchi che l'Italia sta vivendo, realizzando un piano di sostegno nei confronti di chi dovrà subire ancora il peso della gestione dell'accoglienza, che vede in prima linea i nostri sindaci i nostri Comuni, soprattutto quelli più piccoli e più decentrati. *(Applausi)*. I sindaci siciliani, per esempio, che devono sopportare la prima ondata, e poi paradossalmente i sindaci del Nord più profondo, quelli dei Comuni più piccoli e più decentrati di montagna. Sindaci e Comuni agli antipodi in Italia, che si ritrovano a dover gestire situazioni ingestibili che innescano intolleranza e insofferenza, laddove intolleranza e insofferenza non è certo la prerogativa di chi abita territori naturalmente generosi. Negli anni scorsi in territori di montagna come il mio, i sindaci dei Comuni delle nostre valli si sono ritrovati a subire situazioni per cui dalla sera alla mattina le prefetture requisivano strutture e locali per trasformarli alla bell'e meglio in centri di prima accoglienza temporanei temporanei (ce ne sono ancora in piena attività) che poi, appunto, sono diventati permanenti, con paesini da cento abitanti che si sono ritrovati ad ospitare cento migranti senza un piano di integrazione. *(Applausi)*.

ovviamente non credo che possiate immaginarlo, perché governare da dietro una scrivania non consente di vedere cosa succede nel Paese reale. far rivivere a territori già disagiati geograficamente ed economicamente ulteriori disagi e per tutelare parimenti le persone immigrate, noi avevamo già chiesto alla Camera e continuiamo a chiedere oggi in Senato al Governo di tenere conto del parere dei sindaci. Nella litania perenne che continuiamo a ripetere, i sindaci e il Parlamento sono la *task force* dimenticata. I sindaci sono la prima linea, conoscono i territori e il loro parere dovrebbe essere tenuto in assoluta considerazione. Ma la prerogativa di questa maggioranza di Governo è una e una sola: non ascoltare chi andrebbe ascoltato, ritrovandosi poi a prendere decisioni surreali e senza senso, addirittura smontando quello che la precedente maggioranza aveva costruito, come se Conte 1 e Conte 2 fossero due Presidenti del Consiglio diversi. Secondo me è un po' triste che per rimanere in maggioranza ci si vendano i principi. Decreto immigrazione ed eccezionalità e urgenza: entrando nel merito del decreto-legge, con questo provvedimento la norma diventa più aperta rende meno respingente accedere. Considerando che non siamo mai riusciti a governare totalmente il fenomeno e che tanti sono i fattori influenti, in particolare per l'immigrazione dal Mediterraneo (si pensi alla Libia divisa in due, ai Paesi africani in piena guerra civile e affamati, al ruolo di tanti Paesi e ai tanti interessi,

E nemmeno si può dire, come in altri casi di spesa, che finiti i soldi finisce la spesa, perché queste sono azioni a rubinetto, come lo sono gran parte delle spese sanitarie. In Italia, per Costituzione, per civiltà e per cultura, non possiamo dire «opero di peritonite i primi dieci e gli altri li lascio morire»; lo stesso vale per i migranti. Quindi, come faremo quando saranno finiti i soldi? È possibile che non abbiate il benché minimo senso pratico, quell'attenzione del buon padre di famiglia che è il requisito minimo di chi amministra e di chi governa la cosa pubblica? Pertanto, nel provvedimento,

Quindi è una norma ideologica e di contrapposizione politica, questo lo capiamo, ma che almeno sia corretta, sia coperta e abbia i requisiti minimi. Non so se posso prendere qualche minuto in più.

perché se continua così saranno gli italiani a voler scappare. Ci basterebbe anche che un momento così prezioso, che saremo costretti a vivere lontani, come il Natale, non veda degli errori macroscopici: chiudere dal 24 al 27, come previsto; poi riaprire dal 28 al 30, poi richiudere dal 31. che siano *boutade* e illazioni giornalistiche, perché altrimenti saremmo alla follia. Rinsavite. Spero che questa maggioranza, se ci sono componenti che decidono di tirare fuori la testa dalla sabbia, rinsavisca e capisca che non è il tempo di un decreto immigrazione e concludo - che il provvedimento in esame aprirà le porte a tutti indistintamente e farà molto male ai migranti che davvero arrivano per necessità. Farà molto male a tutti perché il vero problema, come ha ricordato prima la collega Binetti, non è solo accogliere, ma integrare.

in questa circostanza, poiché c'è la logica del pacchetto (per cui bisogna votare la fiducia per approvare il provvedimento, poiché in Senato non è possibile fare diversamente), io voterò la fiducia.

effettivamente, da quello che abbiamo sentito oggi, tra inattinenze e *cabaret* di basso livello, a parte qualche intervento, non si è in sostanza parlato del provvedimento. Lo scenario dipinto non è quello reale.

Quindi, quell'equazione salviniana - meno partenze, meno morti - è falsa. Il testo oggi al nostro esame va nella direzione giusta ed è questo il motivo per cui mi violento e voterò la fiducia a questo Governo. Nonostante alcune timidezze, limiti e contraddizioni, il decreto-legge del Governo è stato migliorato nettamente alla Camera dei deputati

si riaffermano criteri di giustizia e principi dello Stato di diritto, ma, nella pratica amministrativa, queste norme consentono anche di rendere più efficienti e meno confusionarie

Come vi dicevo, colleghi del MoVimento 5 Stelle, certamente quei decreti hanno creato condizioni di maggiore insicurezza, come era facile prevedere (non ci voleva, come si dice a Napoli, l'arca di scienza, era immediato). È chiaro che le persone marginalizzate non potessero far altro, nell'irregolarità, che trovare sfruttatori e rivolgersi alla criminalità. Lo dicevamo due anni fa. Benvenuti.

Questo è importante: realizzare in Parlamento qualcosa che abbia finalità che possiamo condividere, senza necessariamente dover inseguire il facile consenso delle masse.

la legge Minniti-Orlando ha cancellato l'appello per una categoria di persone, ovvero ha stabilito che, per alcune categorie, non ci fosse il secondo grado.

come oggi sono da rimuovere alcune storture create dai decreti Salvini. Bisogna però avere il coraggio di andare avanti e di affrontare i problemi ancora esistenti, come diceva la collega Nugnes, in tema di cittadinanza e di giustizia. Nel provvedimento in esame ci sono anche novità importanti, che comunque ci consentono di ripristinare almeno il modesto livello di civiltà *ante* decreto Salvini. Era già modesto, ma vediamo alcuni di questi aspetti. Intanto i permessi di soggiorno possono essere convertiti in permessi di lavoro e questo è importante,

voglio evidenziare che il lavoro parlamentare non è privo di significato, quando è fatto bene e i colleghi della Camera dei deputati hanno fatto un buon lavoro, tutto sommato. Il raccordo tra l'articolo 5, comma 6, e l'articolo 19 evita confusione e discrezionalità da parte dell'amministrazione, stabilendo che può essere rilasciato il permesso di soggiorno per protezione speciale. La propaganda della Lega aveva creato un assetto confuso e un'enorme massa di irregolarità. Il ripristino dell'accoglienza da parte dei Comuni, con gli ex SPRAR, che oggi si chiamano SAI e cioè sistemi di accoglienza integrata per i richiedenti asilo non distingue più, non marginalizza più e quindi non criminalizza i richiedenti asilo rispetto ai titolari di protezione, e questo è un altro dato importante. Finalmente si riapre la possibilità di ingresso per lavoro, con la programmazione e i decreti flussi, da anni bloccati. È dunque importante dire che dappertutto, nel Paese, in quest'Aula, alla Camera

Per entrare in Italia - siamo tutti d'accordo su questo e l'ho sentito da tutte le parti - gli stranieri non si devono rivolgere alla malavita o al trafficante, ma allo Stato, o al trafficante, ma allo Stato, il quale deve avere dei percorsi di accoglienza e di integrazione, come giustamente dicevano alcuni colleghi. affidarsi a delle norme cieche, di chiusura, senza visione e prospettiva, come erano le norme dei decreti Salvini, perché creare un muro in mezzo al mare non ferma il mare, lo devia e quindi arrivano in via autonoma, non ne conosciamo il nome e la storia e non abbiamo sicurezza. Ecco la congiunzione tra immigrazione e sicurezza. ci sarebbero tante cose da dire. Sul decreto sicurezza *bis* qualche passo ancora andava fatto, ma lo tralascio. Per fortuna è stato espunto quel richiamo all'articolo 19 della Convenzione di Montego Bay, perché era sbagliato. Vanno richiamate tutte le Convenzioni e *in toto*, cioè va detto che, nel momento in cui c'è un soccorso in mare, quelle persone non sono più immigrati, ma sono naufraghi e cambia lo *status*. Deve concludere, senatore, mi dispiace. che io sia stato oggetto di espulsione da quel Gruppo politico e oggi non ci sia nemmeno una chiara ammissione di errore da parte loro, non nei miei confronti,

Aspettavo, mi auguravo, auspicavo qualche risposta agli interrogativi che avevo posto, in particolar modo a due interrogativi. Il primo è relativo relativo ai confini: ogni Nazione, ogni Stato, ogni Paese ha una sua specificità, che non è solamente quella del popolo che lo abita, delle leggi che vengono applicate, della moneta, ma ha confini

dai vertici europei per la politica che l'Italia sta adottando. Una politica di apertura, una politica che sta dimostrando di non realizzare davvero nulla di buono, se è vero, come è vero,

alla Guardia di finanza, anche alla polizia municipale; ringrazio tutti coloro che, in buona sostanza, vivono sul territorio il dramma terribile della criminalità. È criminalità ed è innegabile, perché, vedete, l'unico distanziamento che vedo di queste forze politiche è quello dalla realtà. *(Applausi)*. È inutile che raccontiamo agli italiani una narrazione diversa rispetto a quella che è, perché se andiamo in qualsiasi periferia di qualsivoglia città, vediamo qual è la situazione reale che si vive, ed è una situazione drammatica. Sono tanti gli italiani che si trovano a doversi confrontare non solamente per ragioni economiche legate alla povertà, in concorrenza magari con chi è aiutato, con chi ha i sussidi, con chi viene messo all'interno di un circuito che può aiutare a sopravvivere e chi, invece, deve, giorno dopo giorno, riuscire in un qualche modo a sbarcare il lunario, a mettere d'accordo il pranzo con la cena. Colleghi, dovevate abolire la povertà, ma mi pare che la povertà sia aumentata. Se guardiamo i dati Istat, ci rendiamo perfettamente conto che sono circa 6 milioni coloro che vivono in Italia in una condizione gravissima.

giovanile; abbiamo la maglia nera in generale per la disoccupazione. E voi dovete spiegare agli italiani - non so come non ci siate ancora riusciti - come mai si parla ancora di quote. Non abbiamo quote sufficienti di stranieri in Italia in questo momento? Questo è un altro elemento che dovrebbe farvi riflettere. Allora, se è così, dovreste anche rendervi conto che il provvedimento è sbagliato. Non stiamo aiutando coloro che arrivano; li stiamo mettendo in condizioni di estremo ed enorme disagio, perché non ci sono le garanzie minime per consentire a costoro di permanere sul territorio nazionale in condizioni di dignità

ricordare che la cittadinanza non è un diritto, ma uno *status.* Se sei cittadino italiano, devi avere delle prerogative, non puoi essere messo in una condizione di minorata sovranità, nel momento in cui domani magari arriva qualcuno e sbarca. Bisogna anche considerare che la spesa annuale, solamente per quella diretta, ammonta a 5 miliardi di euro.

diminuiranno le entrate tributarie, aumenteranno i licenziamenti e in tutto questo quadro non avete ancora spiegato agli italiani come mai dite che debbano ancora continuare ad arrivare stranieri, non si capisce per cosa. Lo abbiamo già chiarito questa mattina, dicendo con grande precisione che siamo d'accordo su un principio: consideriamo il razzismo un'infezione dello spirito, ma al tempo stesso lo consideriamo anche nei confronti degli italiani, degli italiani, soprattutto nel momento in cui si applicano principi alla rovescia, cioè gli italiani hanno i doveri e coloro che arrivano in Italia hanno tutti i diritti. Questo infatti si verifica, perché, nel momento stesso in cui

Allora cosa andate a raccontare? Cosa dite al vostro elettorato? In particolare mi riferisco alle sinistre, perché in quest'Aula ne abbiamo due. Abbiamo la sinistra dei 5 Stelle, che mi appare in una condizione politica bipolare, perché, se ci mettessimo in sintonia con quello che raccontavano un anno fa sugli stessi provvedimenti e se andassimo a leggere gli interventi o a ricordare

È solamente la volontà di mantenere in piedi questo Governo? Mi rivolgo anche alla sinistra del Partito Democratico, quella che avrebbe dovuto difendere gli interessi degli umili, degli ultimi. Penso alle sinistre che si sono sempre battute per aiutare coloro che trovano enorme difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena, i disoccupati, gli emarginati. Cosa andiamo a raccontare, nel momento stesso in cui

abbiamo valutato ciò che si doveva realizzare in termini di legislazione, e abbiamo riscontrato in quella australiana una superiorità rispetto alle altre. Ad esempio, il Giappone ha un'immigrazione sostanzialmente pari a zero;

un tipo di immigrazione più o meno analogo a quello del Canada, dove viene valutata soprattutto la capacità degli immigrati di realizzare un'attività.

cui noi potremo mettere fine a questa legislazione e a questi principi, che vanno contro l'Italia e soprattutto contro gli italiani. Queste sono le ragioni per le quali voteremo no e daremo tutto il nostro apporto in futuro, affinché possano essere abrogate le leggi che non aiutano il popolo italiano, perché meritiamo davvero, in un momento difficile come questo, una sorte diversa.

e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale; premesso che: ai